presidio della competitività, della produzione e del mantenimento dei livelli occupazionali dello stabilimento ex Sevel di Atessa, sottolineo che l'azione del Governo sin dal relativo insediamento è andata, e prosegue tuttora, nella direzione sollecitata dai senatori interroganti, in una prospettiva tuttavia complessiva, che intende fronteggiare le evidenti problematiche, ma anche valorizzare le opportunità dell'intero comparto *automotive* italiano. Il Mimit ha promosso un confronto continuo, dinamico e costruttivo con gli *stakeholder* del comparto *automotive* e con le altre amministrazioni competenti, che ha condotto anche all'apertura di un tavolo dedicato, muovendosi nella convinzione della relativa rilevanza strategica per il tessuto industriale del Paese, ma anche della necessità di un rilancio della produzione italiana che negli ultimi anni ha conosciuto una costante contrazione e che ora deve affrontare le sfide industriali e ambientali poste da un contesto europeo e internazionale in piena evoluzione. In primo luogo, è stato recuperato rispetto al passato un dialogo costante e positivo con Stellantis. Si sta analizzando la situazione, stabilimento per stabilimento, valutando le prospettive e le migliori soluzioni possibili. In particolare, il confronto riguarda il piano industriale dell'azienda in Italia e all'estero e i temi dello sviluppo, del rilancio e della salvaguardia dei livelli occupazionali. Come è stato ribadito anche dal ministro Urso, il Governo si è posto l'obiettivo di coordinare gli sforzi e le risorse su diversi livelli e diversi fronti in modo sinergico e organico, mirando a favorire le migliori condizioni infrastrutturali, strutturali e di mercato adatte a stimolare la ricerca, lo sviluppo e l'attrazione degli investimenti per mantenere la produzione in Italia. Il confronto intrapreso porterà a un piano di lavoro condiviso al fine di migliorare la competitività e la produttività del settore *automotive.* Con riferimento alla Sevel di Atessa, Sellantis ha confermato il ruolo di *leadership* dell'azienda nella *businnes* *unit* dei veicoli commerciali con la piattaforma di Ducato, ampliando la produzione con il *brand* Opel e con l'accordo per la produzione di veicoli commerciali Toyota. L'impegno del Governo avverrà, dunque, garantendo la più stretta condivisione degli obiettivi con le parti coinvolte, nonché il monitoraggio degli sviluppi

dopo essere stata sequestrata, è stata riaperta con una procedura semplificata. Tutte le discussioni e le mozioni, anche quella che abbiamo approvato ieri, appaiono impotenti perché sono impotenti. Oggi, ironia della sorte, inizia il processo su quello che è accaduto tre anni fa, per cui al danno la beffa: è beffata la giustizia, sono beffati i messaggi del Presidente della Repubblica, è beffato questo luogo che dovrebbe stabilire la regola dello Stato, ma la regola nel mondo del lavoro non è sopravvivere, ma appare morire se, nella stessa azienda, dopo tre anni accade che tre persone muoiano morte altre tre. Formazione, sicurezza, cultura della sicurezza: senza dubbio dobbiamo investire, ma dobbiamo interrogarci sul fatto che questi accadimenti uccidono la credibilità di tutte le istituzioni. Accompagnare i cittadini, difenderli e tutelarli sul luogo del lavoro: anche di questo parliamo quando affrontiamo il tema della ex Sevel, oggi FCA Italy. Stiamo parlando del sito produttivo più importante della Regione Abruzzo e di uno dei più importanti d'Italia e del mondo dell'*automotive*.

lavoratrici e lavoratori e che in poco tempo ha perso 1.000 lavoratori che non sono stati confermati; uno stabilimento che passa da una capacità produttiva di 350.000 furgoni a 250.000 furgoni; uno stabilimento che sta incentivando l'esodo, di cui non si capisce la prospettiva, se non quella di avere investito in una delocalizzazione in un Paese che giustamente anche nei processi di transizione digitale ed ecologica e poi non mette alcun vincolo rispetto alla possibilità che a un certo punto decidano di investire fuori.

parliamo di migliaia di altri posti di lavoro dell'indotto; un indotto complesso, anch'esso non accompagnato nei processi di transizione. Allora, di fronte a quello che sta accadendo, anche rispetto alle mutazioni dell'economia, questo Paese questo Paese deve decidere di avere una politica industriale, perché vanno bene i tavoli, vanno bene i confronti, ma non va bene farsi portare in giro dal *management,* farsi raccontare che senza dubbio si investirà, si manterrà, si svilupperà e allo stesso tempo però succede altro. In quel luogo, allo stato attuale, anche se lei dice che Stellantis ha parlato di salvaguardia dei posti di lavoro e di rilancio, non c'è né salvaguardia né rilancio. C'è bisogno di riflettere davvero su qual è la strategia del nostro Paese in questo settore - è vero - sito per sito, ma definendo esattamente cosa accade, anche con trasparenza e chiarezza nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori

in un territorio che su questo ha costruito un pezzo del suo passato, il presente e vuole investire sul futuro. Senza dubbio la situazione è complessa. Senza dubbio siamo sfidati da quello che ci accade intorno, dai processi di ridefinizione geopolitica anche nel mondo del lavoro, dalle transizioni. Tuttavia, senza una politica, senza chiarezza, senza avere la schiena dritta anche nelle relazioni tra Stato, territorio e attività

made in Italy*. Signor Presidente, il tema sollevato è stato trattato dal Ministero delle imprese e del *made in Italy* nel corso dell'audizione al Senato sulle linee programmatiche lo scorso gennaio 2023. Come correttamente rileva il senatore interrogante, la normativa nazionale ha determinato limiti di campo elettromagnetico più stringenti rispetto a quanto previsto nella raccomandazione della Commissione europea 1999 CE e delle relative applicazioni negli Stati membri, ovvero 6 volt/metro rispetto a 61 volt/metro previsti dalla normativa europea di settore. Peraltro, la raccomandazione a sua volta è stata emanata in recepimento dei risultati delle ricerche scientifiche esposti nelle linee guida redatte dalla Commissione internazionale per la protezione dalle radiazioni non ionizzanti e per la protezione della popolazione dall'esposizione ai campi elettromagnetici, magnetici ed elettrici. In particolare, la legge quadro sulla protezione dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (la legge n. 36 del 2001) è fondata sul principio di precauzione e attribuisce allo Stato le funzioni relative alla determinazione dei limiti di esposizione dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, con lo scopo di dettare criteri unitari e normative omogenee, anche al fine di tutelare l'ambiente, la salute e il paesaggio. Questa determinazione è stata effettuata con il DPCM 8 luglio 2003, richiamato dal senatore interrogante, anch'esso più restrittivo della raccomandazione di cui sopra, in base al principio di precauzione. Su tale tematica è stato sentito il Ministero della salute, il quale ha ribadito che i valori fissati dal citato DPCM 8 luglio 2003 rappresentano una misura di cautela nei confronti di effetti che sono ancora definiti possibili, in quanto non ancora dimostrati dalle attuali conoscenze scientifiche. Nonostante non si trovi supporto nella letteratura scientifica nello stabilire un limite certo e definito all'esposizione a tali campi per la prevenzione di effetti dannosi per la salute, l'impianto normativo italiano vigente, con la definizione dei valori di attenzione, si prefigge di garantire al meglio la tutela della salute umana, avendo l'obiettivo di minimizzare in via precauzionale l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici. Pertanto si terrà conto delle suesposte considerazioni per una revisione della normativa che miri a sviluppare velocemente ed efficacemente i servizi 5G per i cittadini e le imprese, contemperando tale esigenza con quelle connesse all'ambiente e alla salute. Nell'attuale contesto di sviluppo tecnologico e di maggiore consapevolezza da parte di tutti della strategicità del digitale e dei reali impatti della tecnologia sulle nostre vite, è possibile un compromesso che bilanci in modo equo gli interessi di tutti gli attori in gioco. Si tratta di un tema molto importante e molto delicato, al quale è dedicato peraltro un apposito tavolo tra tutte le amministrazioni coinvolte, presieduto proprio dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il Mimit ha da tempo proposto una riflessione sulla peculiare restrizione cui sono vincolati gli operatori italiani rispetto ai *competitor* europei, pur avendo sempre come riferimento la salvaguardia della salute dei cittadini, e ha a tal fine, tra l'altro, commissionato un apposito studio sul tema in parola, a valle del quale potranno essere valutati opportuni interventi anche di tipo normativo.

In questa fase e nell'attuale congiuntura particolarmente difficile le infrastrutture digitali stanno diventando sempre più un reale alleato di chi fa impresa, di chi crea valore sul territorio.

restrittivi rispetto al mercato europeo. La raccomandazione europea, che è stata recepita da altri Stati importanti quanto l'Italia, come Francia, Spagna e Germania, fa sì che altri Stati possano correre più velocemente e le imprese essere più competitive rispetto a quella della nostra Nazione. È vero che il Ministero della salute ha detto che non ci sono ad oggi studi scientifici in merito; ma è altrettanto vero che la comunità scientifica europea ha autorizzato

possa garantire anche l'Italia per rilanciare e portare i limiti - come diceva prima il Sottosegretario - a un adeguamento verso l'alto per il mondo delle telco, che hanno valutato il *gap* tecnico di copertura nazionale in un mancato ritorno che si aggira tra i 2,9 e i 4,3 miliardi. Ciò vuol dire possibile mancanza di gettito per lo Stato, ma anche valore e indotto per le imprese italiane in un mercato sempre altamente competitivo come quello europeo e internazionale.

questa Nazione si è posta nel progetto del PNRR e, quindi, è fondamentale raggiungere detti obiettivi. È sempre all'ordine del giorno in quest'Aula e allo stesso tempo a Montecitorio che gli obiettivi del PNRR per noi per il nostro sistema Paese debbano essere raggiunti. Quindi, accolgo con soddisfazione l'apertura del Ministero e mi auguro che quanto prima questo provvedimento normativo venga approvato per il bene della nostra Nazione e di chi fa impresa, che è sempre in prima linea. finestra") sull'operatività degli stabilimenti di raffinazione ISAB, in provincia di Siracusa. l'interrogazione in parola ripercorrere le diverse iniziative, anche normative, adottate dal Governo per la salvaguardia dello stabilimento ISAB e del relativo indotto operante nel polo petrolchimico di Priolo Gargallo (Siracusa), a fronte delle ripercussioni della crisi ucraina, in particolare connesse alla previsione di embargo all'importazione del petrolio russo a partire dal 5 dicembre 2022. Al riguardo, rappresento che ISAB è una realtà di primaria importanza per il settore energetico e per il territorio in cui è inserita. Nella decisa volontà di salvaguardare una realtà tanto strategica per l'economia nazionale, la reazione del Governo dinanzi alla contingenza eccezionale indotta dalla crisi ucraina è stata celere e aperta a percorrere strade differenti, per approdare poi alla soluzione valutata più efficace e idonea. In tale direzione è intervenuto *in primis* il decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, convertito poi in legge il 30 gennaio 2023, richiamato dal senatore interrogante e con il quale sono state previste specifiche misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi

Nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono altresì riconosciuti beni strumentali allo stabilimento industriale gli impianti di depurazione di Priolo Gargallo e Melilli, perché infrastrutture necessarie ad assicurare la continuità produttiva dello stabilimento. Frattanto è proseguita ed è andata a buon fine la trattativa per la vendita dello stabilimento di Priolo al fondo di *private equity* GOI Energy con sede a Cipro, che ha portato all'attuale assetto proprietario. In questo contesto, il Mimit ha seguito la trattativa ed è stata avviata una dettagliata istruttoria per accompagnare la cessione degli impianti con esercizio dei poteri speciali previsti dalla normativa sul *golden power* (articolo 2 del decreto-legge 15 L'operazione è stata autorizzata subordinatamente al rispetto di una serie di prescrizioni richiamate anche dal senatore interrogante, interrogante, volte a garantire, tra l'altro, la continuità delle forniture, della produzione e dei livelli occupazionali, nonché la disponibilità degli investimenti necessari all'attuazione del piano di transizione verde nell'ambito di un più ampio piano industriale di medio e lungo periodo che dovrà essere certificato in maniera indipendente da un soggetto terzo. L'intervento del Governo, quindi, è stato tempestivo, determinante e anche congruo nel muovere verso la tutela della sicurezza energetica e del lavoro. In prospettiva, si proseguirà nel confronto tra i diversi attori coinvolti e si monitoreranno gli sviluppi della decisione assunta. Già lo scorso 23 maggio, presso il Mimit, si è tenuto un incontro al quale hanno partecipato il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero dell'economia delle finanze, i rappresentanti del territorio e le organizzazioni sindacali. Nel corso dell'incontro è stata ribadita la volontà di adoperarsi affinché sia data completa attuazione alle misure contenute nel DPCM del 3 febbraio 23, che prevedono per Priolo il bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione con quelle di tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute e dell'ambiente. Resta fermo, dunque, l'impegno del Governo ad adottare, ove tali impegni non siano mantenuti, tutte le iniziative ritenute necessarie.

febbraio 2023 e chiedeva, tra le altre cose, quali fossero le garanzie, dal punto di vista degli investimenti, di un piano industriale di lungo periodo di transizione ecologica in quella zona, cioè quali sono le caratteristiche che fanno sì che ci sia un piano industriale di medio-lungo periodo agganciato a REPower EU, ai fondi europei; e chiedeva quali fossero le misure aggiuntive rispetto ai titoli che sono stati riportati nella sintesi del DPCM attuato in applicazione delle prescrizioni del *golden power.* Chiedevamo, inoltre, di sapere quali fossero i meccanismi che garantissero la stabilità occupazionale in un contesto nel quale l'impegno di permanenza dell'acquirente è solo di cinque anni rispetto a un piano industriale di medio-lungo periodo. Nello stesso tempo, visto che persistono le ragioni di natura geopolitica che hanno indotto il decreto alla possibile introduzione di una

tale previsione non sia stata applicata. E lo chiedevamo in considerazione del fatto che qui abbiamo avuto semplicemente un passaggio di proprietà, ma non una cessazione delle cause che hanno portato il Governo a realizzare il primo decreto, quello cioè che ha stabilito la possibilità di avere un meccanismo di intervento temporaneo da parte del pubblico. Non posso che essere contento del fatto che nell'incontro del 23 maggio - come ci è stato riferito - si sia ribadita la volontà di andare avanti su queste misure,

proprio nell'impianto, ha ribadito la sua volontà, che noi apprezziamo molto, di fare di tutta quella zona industriale un *hub* energetico nel Mediterraneo. Vorrei sapere

Tali prescrizioni, almeno dalle notizie di stampe che noi abbiamo potuto verificare, sono talmente generiche da non prefigurare degli impegni precisi verificabili, soprattutto con un sistema di *enforcement* che garantisca quegli obiettivi. Si tratta come lei ha ricordato - di una realtà che ha un indotto complessivo che coinvolge almeno 3.000 occupati, diverse imprese dell'indotto, rappresentando una quota significativa dell'esportazione di prodotti raffinati dall'Italia e soprattutto un fabbisogno di oltre il 40 per cento, soddisfatto da quel tipo di zona industriale sulla raffinazione italiana. Tutte queste cose messe insieme fanno capire che ha fatto bene - e noi abbiamo condiviso - il Governo a intervenire, ma quel tipo di intervento poi, nei fatti, non si è ancora manifestato. Rinnovo qui a lei e lo faremo nuovamente con atti di sindacato ispettivo la richiesta di avere informazioni più dettagliate sulla tempistica e soprattutto sulle garanzie che il piano industriale di medio e lungo periodo e quello occupazionale siano coerenti tra di loro in termini di durata temporale, ma soprattutto che vi sia la prospettiva seria di una forte capacità di investimento nella transizione ecologica ed energetica, che è il punto di svolta che tutti i lavoratori e le imprese si attendono

Le disposizioni introdotte dal Governo per far fronte all'eccezionale aumento dei prezzi dei materiali da costruzione prevedono la possibilità per le stazioni appaltanti di accedere a fondi appositamente istituiti presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In relazione alle attività di erogazione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1-*septies*, comma 8, del decreto-legge n. 73 del 2021, relativo alla compensazione dei prezzi per le lavorazioni eseguite nel secondo semestre dell'anno 2021, il MIT ha ripreso l'*iter* volto all'erogazione dell'acconto del 50 per cento a inizio dello scorso mese di maggio. Tale procedura era stata sospesa a settembre 2022 a causa di un contenzioso, conclusosi favorevolmente con sentenza TAR-Lazio n. 6984 del 19 aprile 2023, citata dall'onorevole Basso. A fine luglio del corrente anno è stata interamente conclusa l'istruttoria relativa all'acconto del 50 con lo stanziamento di circa 51 milioni di euro a favore di tutti gli enti beneficiari. Il relativo decreto ministeriale n. 171 del 9 agosto scorso ha approvato la ripartizione delle risorse del fondo in piccola, media e grande impresa ed è attualmente al vaglio della Corte dei conti. In riferimento all'attualità 2022 circa le attività di erogazione delle risorse del fondo di cui all'articolo 26, comma 4, lettera *a)*, del decreto-legge quanto al primo semestre sono state concluse le attività istruttorie di tutte le istanze presentate. Sono state ammesse a contributo 681 istanze e attribuite risorse per un importo complessivo pari a circa 74 milioni di euro. In merito al secondo semestre, sono state concluse le attività istruttorie e ammesse a contributo 577 istanze, per un importo complessivo pari a circa 138 milioni di euro.

(MIT) ha proceduto all'accertamento dei presupposti minimi delle oltre 2.000 richieste di accesso al fondo e nel corrente mese di settembre è stato già erogato l'acconto del 50 pari a 229 milioni di euro a favore di circa il 99 per cento degli enti beneficiari. Ad oggi, è in corso di predisposizione il decreto di ripartizione delle risorse del fondo in piccola, media e grande impresa, ai fini dell'erogazione del saldo. In merito al secondo semestre, è in corso l'accertamento dei presupposti minimi per l'accesso al fondo delle oltre 1.700 richieste pervenute, per un valore complessivo di circa 560 milioni di euro. Per quanto attiene alle iniziative del MIT per accelerare le procedure di pagamento, tra le misure messe in campo negli ultimi mesi ricordo che il comma 458 della legge di bilancio 2023 ha unito in un unico fondo le richiamate procedure di cui alle lettere introducendo i commi 6-*bis* e 6-*ter* al citato articolo 26 del decreto-legge n. 50 del 2022. Il relativo decreto ministeriale di attuazione ha inoltre aumentato le finestre temporali per la presentazione delle istanze, passando dalle precedenti due alle attuali quattro, ovvero aprile, luglio e ottobre 2023 e gennaio 2024, disponendo l'immediata lavorazione nel mese successivo. Infatti, relativamente alla scadenza della prima finestra temporale del 30 aprile 2023, sono state tempestivamente concluse le attività istruttorie entro il 31 maggio e ammesse a contributo 1.585 istanze, per un importo complessivo pari a circa 245 milioni di euro. Il decreto di ammissione a fondo è stato registrato alla Corte dei conti il 22 giugno scorso e il successivo 27 giugno sono stati emessi il decreto dirigenziale di impegno e liquidazione e relativi ordini di pagamento. Anche relativamente alla scadenza della seconda finestra temporale del 31 luglio, sono state tempestivamente concluse le attività istruttorie e ammesse a contributo 2.913 istanze, per un importo complessivo di oltre 458 milioni di euro. Il relativo decreto, il n. 190 dell'8 settembre scorso, è all'esame degli organi di controllo. Inoltre - come riportato dal senatore Manca - presso il MIT è stata attivata un'apposita *task force* per consentire un'accelerazione della lavorazione delle istanze pregresse nonché delle nuove, anche alla luce dell'aumento delle finestre temporali. Infine, l'articolo 11 del decreto-legge n. 75 del giugno 2023 ha introdotto una ulteriore semplificazione delle procedure con la previsione di controlli a campione sulle istanze di accesso al fondo. Tali iniziative testimoniano l'impegno del Ministero per scongiurare qualsivoglia previsione negativa sui tempi per il completamento dei pagamenti e per accelerare le procedure a favore delle imprese e dei lavoratori.

la risposta, ma vorrei riprendere due considerazioni aggiuntive, che collocano un po' nell'attualità

e sappiamo bene - è una regola dell'economia, non dipende dal colore politico del Governo - che, di fronte a tassi di interesse crescenti, se si bloccano gli investimenti si spinge l'Italia in recessione.

Ci sono tre miliardi di euro destinati ad affrontare una questione che riteniamo cruciale e che, di fronte a tassi di interesse crescenti, non può consentire al Governo di trattenere risorse nel bilancio dello Stato, quando si tratta di liquidità essenziale per evitare non solo il blocco dei cantieri, ma io dico anche il fallimento di numerose imprese che, dovendo ricorrere al credito con tassi di interesse così alti, non avrebbero le condizioni per reggere non solo la realizzazione di quell'appalto, ma il sostegno al lavoro, alla crescita e allo sviluppo economico del nostro Paese. Quindi, la considerazione che facciamo è molto semplice: non possiamo permetterci, di fronte a questo quadro economico, che il Paese rallenti il processo di investimento pubblico e privato.

e se, a questo punto, anche le opere cosiddette minori, non oggetto di finanziamento, non trovano nella liquidità a disposizione del Governo una risposta immediata, questo Paese lo si spinge certamente in recessione. Questa è una responsabilità politica grave, che il Governo non può permettersi. Mi auguro che, anche di fronte all'ormai imminente nota d'aggiornamento al DEF, ma soprattutto con la legge di bilancio, si compiano tutti gli sforzi per evitare che liquidità e fondi già destinati impieghino così tanto tempo per arrivare alle imprese e alle stazioni appaltanti. In questo momento, infatti, sono più le opere bloccate per l'incapacità di produrre una revisione dei prezzi, peraltro coperta da questi fondi, che quelle che riescono a completare l'*iter* e quindi a velocizzare la realizzazione e la conclusione di lavori fondamentali, non solo per le singole comunità, ma per l'intero Paese. Sappiamo tutti che, senza investimenti pubblici e privati, questo Paese lo spingerete in recessione e ne porterete una responsabilità politica, che riteniamo molto importante. Qui stanno a zero le chiacchiere e sta a zero l'opposizione al passato. Ci sono le risorse: invece di parlare di propaganda, si facciano azioni concrete e si metta nelle condizioni il Governo di governare invece di parlare senza velocizzare gli investimenti pubblici e privati, che saranno essenziali per il futuro del nostro Paese.

In merito all'atto di sindacato ispettivo, ringrazio l'onorevole senatore per aver portato all'attenzione di questa Assemblea un tema così importante, quale l'ammodernamento di una importante infrastruttura viaria come la E45. Al riguardo, la società Anas ha rappresentato quanto segue. I lavori in corso sull'itinerario E45-E55 rientrano in un vasto programma di manutenzione straordinaria per la riqualificazione dell'itinerario Orte-Mestre. Dette attività riguardano, tra l'altro, il risanamento di ponti e viadotti, l'ammodernamento delle barriere di sicurezza, la realizzazione della *smart road*, il rifacimento della segnaletica e il risanamento profondo della pavimentazione. Tali interventi garantiranno un sensibile miglioramento del livello di servizio e delle condizioni di sicurezza della strada. Con riguardo alla sola E45, sul tratto umbro, in prossimità dello svincolo di Montone, sono in corso lavori di risanamento strutturale dei viadotti Tevere 1 e Tevere 2, che prevedono la parziale demolizione e ricostruzione dell'impalcato, l'installazione di dispositivi di appoggio antisismici e il risanamento dei calcestruzzi. Il completamento dei lavori è previsto entro il corrente anno. Per quanto attiene al tratto emiliano-romagnolo tra Verghereto e Cesena sono attivi 14 interventi, in particolare lungo l'intero tracciato della strada statale 3-*bis* Tiberina, dallo svincolo di Canili allo svincolo di Cesena Nord. Sono attualmente in corso sei attività di manutenzione straordinaria su ponti e viadotti. Tra le principali segnalo quelle relative al viadotto Teverola 2, al chilometro 164,300, la cui ultimazione è prevista entro la fine del corrente mese.

l'ultimazione per il mese di marzo 2024. Per quanto attiene alle gallerie, sono attualmente in corso tre interventi per ripristini strutturali e per l'adeguamento degli impianti tecnologici. Il principale riguarda la galleria lago di Quarto al chilometro 190. Le attività di cantiere stanno interessando attualmente la canna in direzione Nord, con ultimazione prevista entro il mese di novembre 2023 successivamente saranno avviate le lavorazioni lungo la canna in direzione Sud, con fine prevista entro il mese di giugno 2024. Tali interventi vengono programmati in modo che le corrispondenti lavorazioni non risultino tra loro interferenti ovvero non determinino restrizioni alla fruibilità dell'infrastruttura che possono penalizzare l'utenza. Per tale motivo attualmente risultano in fermo cantiere quelli afferenti all'installazione di barriere di spartitraffico e quelli concernenti il ripristino strutturale e l'adeguamento degli impianti tecnologici in direzione Sud della galleria Verghereto al chilometro 167,400. Tali opere di manutenzione e di ammodernamento rappresentano una priorità per garantire la mobilità dei cittadini e favorire la vocazione turistica e imprenditoriale di questa importante arteria stradale. In riferimento al rispetto del cronoprogramma, il MIT monitorerà la continuità operativa dei cantieri e ha interessato Anas affinché venga assicurata la conclusione dei lavori nei tempi previsti.

tuttavia, non posso dichiararmi soddisfatto perché i quesiti che ponevamo con l'interrogazione erano diversi. Conoscevamo più o meno gli stanziamenti e gli appalti che Anas ha messo in essere da qualche tempo, anche perché, senza prendere meriti di parte, tutte le forze politiche, tutti i Comuni e tutte le Regioni interessate da questa importante arteria negli anni scorsi si sono battuti per poter cominciare a ripristinare un minimo di sicurezza e di decoro in quella che in certi tratti - non è un'esagerazione - era diventata una mulattiera per molti motivi. Qualche errore di progettazione decenni fa? Possibile. Problematiche nate, specialmente nella zona di Verghereto, qualità del terreno, che peraltro è vicino al corso del Tevere appena nato dal monte Fumaiolo? Possibile. Sta di fatto che

da quasi tutte le forze politiche, quindi i lavori sono un merito di tutti e delle istituzioni locali. Tuttavia questi lavori, signora Sottosegretaria, vanno clamorosamente a rilento. Io sono un utente di quella strada, la percorrono due o tre volte la settimana da Città di Castello fino a Orte, proprio lo scorso fine settimana ero a Ravenna, quindi è

quando anche in epoche passate, per tratti di strade e su sollecitazioni anche nostre, Anas aveva lavorato per dare continuità ai lavori, lavorando sette giorni su sette,

quindi la E45, che poi diventa E55 da Cesena a Ravenna, è fondamentale, non solo per gli umbri pendolari, ma per tutti coloro che da Roma vogliono andare a Bologna senza passare per Firenze, perché anche la Variante di di Valico - benemerita, per carità - presenta, come noto, quotidianamente delle criticità, soprattutto tra Firenze e Prato, con chilometri e chilometri quotidiani di fila. Pertanto questa arteria è è un'alternativa importante; se - Dio non voglia - si bloccasse l'autostrada del sole, è evidente che la E45 diventerebbe un'alternativa fondamentale.

creando problematiche e incidenti. Abbiamo sollecitato Anas anche su questo, chiedendo di mettere barriere e reticolati per ridurre al minimo questo rischio; sembra una cosa marginale, ma non lo è in quelle realtà, perché cinghiali, caprioli e altri animali sono anche questi aspetti di vita quotidiana, su cui francamente vedo troppa disattenzione.

rappresento preliminarmente che l'attività di predisposizione dei decreti attuativi della legge n. 99 del 2022 costituisce una priorità del Ministero dell'istruzione e del merito, il quale, fin dall'insediamento di questa compagine di Governo, ha dedicato particolare impegno anche organizzativo a questo scopo, procedendo secondo un preciso cronoprogramma e un metodo di lavoro che si è svolto in maniera concertata con le Regioni. Ricordo, infatti, che l'ordine di priorità di tali decreti attuativi e le principali linee di indirizzo degli stessi sono stati condivisi con le Regioni nell'ambito di un intenso confronto preliminare con le stesse, il quale sta proseguendo adesso nel merito dei singoli provvedimenti. Questa impostazione di lavoro ci ha consentito di concludere già l'*iter* comprensivo della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* di tali decreti ministeriali, concernenti le seguenti tematiche: costituzione e funzionamento del comitato nazionale ITS Academy, costituzione delle commissioni delle prove di verifica finale delle competenze acquisite relativa certificazione, nonché modelli di diploma di specializzazione e definizione dello schema di statuto delle fondazioni ITS Academy. A ciò aggiungo che vi sono altrettanti decreti attuativi in fase di istruttoria avanzata, prossimi all'approvazione e all'entrata in vigore. Mi riferisco in particolare al decreto in tema di riconoscimento e accreditamento degli ITS Academy, sul quale è stata acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano. Il medesimo decreto è stato trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti per l'acquisizione del prescritto parere, calendarizzato proprio in questa settimana. Ottenuto il parere, il testo potrà essere sottoposto alla firma del Ministro e inviato ai competenti organi di controllo. In merito al decreto recante «Disposizioni concernenti le aree tecnologiche e le figure professionali nazionali di riferimento degli ITS Academy», evidenzio che, a seguito di approfondita interlocuzione in appositi tavoli tecnici con le parti interessate, si è addivenuti a un testo condiviso, che ha ottenuto il parere favorevole del Consiglio superiore

Segnalo che il decreto è stato trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti per l'acquisizione del parere, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 99 del 2022. Successivamente anch'esso potrà essere sottoposto alla firma del Ministro. Infine segnalo che il terzo decreto, che definisce i criteri per autorizzare un ITS Academy ad operare in una o più aree tecnologiche, ha già ricevuto il parere favorevole del Consiglio superiore della pubblica istruzione ed è dunque ormai prossimo alla sua adozione. Concludo assicurando che per i restanti provvedimenti attuativi il Ministero procederà con il medesimo metodo fin qui seguito, continuando ad operare nel rispetto del principio di leale collaborazione e a mantenere un proficuo e costante confronto con le Regioni e le fondazioni ITS Academy. Solo grazie a questo metodo di continuo e reale confronto con le citate istituzioni, infatti, si renderà possibile continuare a conseguire i risultati dinanzi illustrati, assicurando il perfezionamento, nei tempi previsti dal PNRR, dei restanti decreti attuativi necessari a definire compiutamente la riforma degli ITS Academy.

fortemente condiviso dal Parlamento, una delle poche riforme passate quasi all'unanimità, a significare la consapevolezza diffusa che questo Paese è la seconda manifattura d'Europa e quindi ha bisogno di colmare un *gap* rispetto ad altri Paesi come Germania e Francia (per fare solo alcuni esempi), per quanto riguarda la carenza di tecnici quindi due bisogni fortemente sentiti dal Paese: da un lato la necessità di non tradire le aspettative dei giovani in termini di realizzazione del proprio talento e della propria competenza, ma anche aspettative occupazionali adeguate, dall'altro lato l'esigenza delle imprese di ottenere quelle professionalità indispensabili per la loro competitività. Per molti anni questo Paese si è diviso attorno al tema delle risorse. Io penso che il tema delle risorse sia stato troppo spesso un alibi, che il Piano nazionale di ripresa e resilienza ha accantonato, stanziando un miliardo e mezzo di risorse sugli ITS. Ora non è pensabile, Sottosegretaria, che, a distanza di tanti mesi, anzi ormai di un anno, dall'approvazione della riforma, dei tredici decreti attuativi indispensabili per misurare l'efficacia e l'operatività di quella riforma ne siano stati completati solo tre o forse quattro. Comprendo che l'*iter* è complicato e che non è solo nelle mani della politica, perché sono spesso anche i responsabili amministrativi all'interno del Ministero dell'istruzione a dover correre. Ma certo senza l'attuazione tempestiva non di tre o quattro decreti, ma dei tredici decreti attuativi, noi rischiamo di rappresentare quella riforma come non efficace, quando in realtà è una riforma meramente approvata dal Parlamento, ma non operativa. Quindi mi affido a lei, conoscendo la sua passione per la scuola e l'educazione in generale, affinché ci sia un'accelerazione: ne abbiamo bisogno anche al fine di spendere nel miglior modo possibile le risorse che il PNRR mette a disposizione, risorse che devono servire non per moltiplicare i posti all'interno delle fondazioni degli ITS, ma per moltiplicare i corsi, alzando l'asticella della qualità. Davvero confido che questi decreti attuativi, che certo devono vedere il coinvolgimento un'assunzione di responsabilità anche da parte della Conferenza Stato-Regioni e di organi che sono chiamati ad esprimere i pareri, non da ultime le Commissioni parlamentari, nell'arco di pochi mesi completino il proprio *iter*. Penso che nell'anno 2023, che l'Europa ha destinato alle competenze, sarebbe il segnale concreto migliore che tutti noi potremmo dare.

Signor Presidente, con riferimento all'atto di sindacato ispettivo indicato, deve essere posto in risalto che in data 22 marzo 2023 si è tenuto l'incontro tra la parte pubblica e le organizzazioni sindacali in merito alla sottoscrizione delle ipotesi di accordo sulle progressioni economiche per l'anno 2022, sui criteri di pagamento del fondo risorse decentrato, relativo all'anno 2020, e sull'*addendum* all'accordo sui criteri di mobilità del personale dell'organizzazione giudiziaria. Alla riunione si è altresì raggiunta un'intesa sui criteri di pagamento del fondo risorse decentrate relativo all'anno 2021. In data 30 maggio 2023 sono stati poi sottoscritti l'accordo sui criteri di pagamento del fondo risorse decentrate relativo all'anno 2020

Alla riunione si è altresì raggiunta un'intesa sui criteri di pagamento del fondo risorse decentrate relativo all'anno 2021. In data 30 maggio 2023 sono stati poi sottoscritti l'accordo sui criteri di pagamento del fondo risorse decentrate relativo all'anno 2020 e l'ipotesi di accordo sui criteri di pagamento del fondo risorse decentrate relativo all'anno 2022. A completamento della procedura si è in attesa dei dovuti controlli da parte del Ministero dell'economia e delle finanze e del Dipartimento della funzione pubblica. È senza dubbio nelle intenzioni di questa amministrazione dare rilevanza alla finalità di incentivare il personale in servizio, attraverso l'erogazione di fondi individuati in modo da garantire elevati *standard* di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, premiando allo stesso tempo il merito. Non sfugge altresì a questo Dicastero, in relazione alle proprie competenze istituzionali, l'urgenza della completa attuazione delle procedure, pure articolate e complesse, prescritte per le progressioni economiche dei dipendenti legittimati. Ciò nella consapevolezza della necessità, da una parte, di riconoscere il giusto valore all'esperienza e alla professionalità maturate e, dall'altra parte, di porre gli uffici giudiziari, come anche le articolazioni dell'amministrazione centrale, nella condizione di avvalersi dell'opera di personale esperto e motivato nell'affrontare carichi di lavoro obiettivamente per assicurare un adeguato servizio giustizia. Nell'atto di sindacato ispettivo viene riportato il resoconto di un'audizione del 2017 del direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, nel corso della quale venivano indicati asseriti risparmi di 63 milioni di euro l'anno per i soli costi riconducibili alle spese sostenute per notifiche e comunicazioni e un presunto risparmio a regime di circa 80 milioni di euro annui. L'articolo 27 del decreto legislativo n. 150 del 2009 prevede che una quota fino al 30 per cento dei risparmi sui costi di funzionamento derivanti da processi di ristrutturazione, riorganizzazione e innovazione all'interno delle è destinata in misura fino a due terzi a premiare, secondo criteri generali definiti dalla contrattazione collettiva integrativa, il personale direttamente e proficuamente coinvolto e per la parte residua ad incrementare le somme disponibili per la contrattazione stessa. Viene espressamente previsto, tuttavia, che le risorse relative a detti risparmi possono essere utilizzate solo se gli stessi sono stati documentati nella relazione di *performance*, validati dall'organismo di valutazione di cui all'articolo 14 e verificati dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. È di tutta evidenza come l'attuazione della norma preveda, quali presupposti concorrenti, che i risparmi siano documentati nella relazione di *performance*, validati dall'Organismo (OIV) e verificati dalla Ragioneria generale dello Stato. Dagli atti e dalle informazioni acquisiti, non risulta se sia verificato alcuno di tali presupposti. Nell'ambito delle relazioni di *performance*, non risulta alcuna dimostrazione o documentazione al riguardo e di conseguenza non sembra aver avuto seguito né alcuna specifica validazione da parte dell'OIV, né la verifica da parte della Ragioneria generale dello Stato. Tale requisito presuppone, peraltro, che il competente direttore generale avrebbe dovuto inserire tali risparmi nell'ambito degli obiettivi di *performance*, dando conto e dimostrazione dell'effettivo conseguimento degli stessi in sede di relazione finale. Inoltre, in occasione della suddetta audizione eventuali risparmi avrebbero potuto essere astrattamente ricondotti alle notifiche in materia civile che, come noto, sono prevalentemente a carico delle parti e di conseguenza i connessi risparmi non possono essere riferiti a risorse del bilancio dello Stato. Al fine di valutare la portata di tale normativa, si ritiene inoltre che vadano contestualmente valutate anche le concorrenti disposizioni previste in materia che, successivamente intervenute, potrebbero essere interpretate in termini di completamento dell'originario quadro normativo. Si fa riferimento, in particolare, all'articolo 15 del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale, come integrato dall'articolo 11, comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235, commi 2-*bis* e e dall'articolo 15, comma 1 del decreto legislativo del 13 dicembre 2017, n. 217, comma 2-*quater*: «2-*bis*. Le pubbliche amministrazioni nella valutazione dei progetti di investimento in materia di innovazione tecnologica tengono conto degli effettivi risparmi derivanti dalla razionalizzazione di cui al comma 2, nonché dei costi e delle economie che ne derivano. 2-*ter*. Le pubbliche amministrazioni, quantificano annualmente, ai sensi dell'articolo 27, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, i risparmi effettivamente conseguiti in attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2. Tali risparmi sono utilizzati, per due terzi secondo quanto previsto dall'articolo 27, comma comma 1, del citato decreto legislativo n. 150 del 2009 e in misura pari ad un terzo per il finanziamento di ulteriori progetti di innovazione. 2-*quater*. AgID individua, nell'ambito delle Linee guida, criteri e modalità di attuazione dei commi 2-*bis* e 2-*ter*, prevedendo che ogni pubblica amministrazione dia conto annualmente delle attività previste dai predetti commi nella relazione sulla gestione di cui all'articolo 11, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118». Si ritiene pertanto che l'intervenuta disposizione, oltre a delineare in maniera più puntuale il quadro normativo con particolare riferimento all'effettività dei risparmi conseguiti, abbiano comportato il superamento della materia *de delle disposizioni previgenti. Dal suo canto, la pubblica amministrazione, nella stessa nota estesa in data 18 luglio 2023, rilevava che il predetto articolo 15 del codice dell'amministrazione digitale stabilisce al comma 2-*quater* che l'AgID individua, nell'ambito delle linee guida, criteri e modalità di attuazione dei commi 2-*bis* e 2-*ter*, prevedendo che ogni pubblica amministrazione dia conto annualmente delle attività previste dai predetti commi nella relazione sulla gestione di cui all'articolo 11, del decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118. Ciò premesso, questa amministrazione, a seguito di accertamenti espletati, avvalendosi della collaborazione del Dipartimento della funzione pubblica, ha appurato di non possedere gli elementi informativi utili. Inoltre, con nota DFP n. 30698 del 10 maggio 2023, è stato chiesto al Ministero dell'economia e delle finanze di fornire informazioni in possesso dello stesso dicastero, acquisite anche in sede di controllo sui contratti integrativi ai sensi dell'articolo 40-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001. In considerazione di quanto previsto dal citato comma 2-*quater* del predetto articolo 15 con nota DFP 30697 del 10 maggio 2023 è stato altresì richiesto

a protocollo DFP 34799 del 29 maggio 2023.

a causa dell'intervenuta disciplina emergenziale legata al contrasto al Covid-19 e all'adozione della modalità lavorativa *smart* *working*, l'attuazione della previsione di quel suddetto articolo 15, comma 2*-quater*, del CAD, non può non tener conto del mutato quadro normativo. Ne deriva che le linee guida previste sono attualmente oggetto di riconsiderazione e completa

Presidente, preso atto del fatto che la normativa, in modo abbastanza chiaro, evidenzia questa premialità e assunto che

ritenuto uno degli elementi cardine, e visto che comunque, come detto adesso dal Sottosegretario, vi è questa premialità dei due terzi, credo che sarebbe veramente utile che si verificasse l'effettività dei risparmi testé richiamati. Sarebbe altresì utile verificare anche la procedura relativa a questo documento di *performance* che, mi sembra di aver compreso dalla complessa risposta all'altrettanto complesso quesito che è stato posto, sottende alla valutazione di questi risparmi stimati che possono essere utilizzati per un fine che tutti tutti noi riteniamo estremamente utile e rilevante ai fini della semplificazione e dell'efficientamento della nostra procedura. Mi riferisco cioè alla valorizzazione del personale, degli amministrativi di giustizia, che hanno una professionalità acquisita, in molti casi, vista anche l'anzianità degli stessi, per il lungo corso e la lunga esperienza da essi esercitata,

ad una progressione, valorizzazione e riqualificazione del personale amministrativo di giustizia che credo sia uno degli elementi cardine per raggiungere la soddisfazione di quella esigenza semplificatoria

Signor Presidente, onorevoli senatori, l'ufficio per il processo è stato previsto dalla legge come una struttura organizzativa finalizzata a garantire la ragionevole durata del processo attraverso l'innovazione dei modelli organizzativi e assicurando un più efficiente impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Si tratta di una struttura tecnica in grado di affiancare il giudice nello svolgimento dei suoi compiti e delle sue attività. All'ufficio per il processo sono invero attribuite tutte le attività di ausilio all'espletamento del lavoro giudiziario, ivi comprese quelle di preparazione e di ricerca necessarie alla risoluzione degli affari e alla stesura dei provvedimenti. Possono essere altresì attribuiti compiti di supporto all'efficiente utilizzo dei sistemi informatici quali, a titolo meramente esemplificativo, il coordinamento e il monitoraggio dei depositi telematici, nonché la tempestiva rilevazione delle problematiche derivanti dall'adozione di nuove tecnologie e di nuovi modelli organizzativi. Piano nazionale di ripresa e resilienza, con riferimento all'investimento M1C1 (capitale umano), ha visto impegnato in maniera assidua l'ufficio per il processo, stante l'importanza dell'obiettivo. In particolare, il decreto-legge del 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'efficienza della giustizia, ha disciplinato le modalità di reclutamento di personale a tempo determinato per il supporto alle linee progettuali per la giustizia del PNRR. Al fine di assicurare la piena operatività dell'ufficio per il processo e di supportare le linee di progetto di competenza del Ministero della giustizia, ha autorizzato, per il periodo 2021-2026 e con contratto di lavoro a tempo determinato, il reclutamento di un contingente massimo di 16.500 unità di addetti all'ufficio per il processo, nonché di 5.410 unità di ulteriore personale amministrativo non dirigenziale in profili specifici di area 2 e area 3, anche tecnici, quali ad esempio edili, contabili e informatici, così ripartiti: 1.660 unità complessive per i profili di area 3, fascia economica F1; 750 unità complessive per i profili di area 2, fascia economica F2; 3.000 unità nel profilo di operatore di *data entry* area 2, fascia economica F1. Le procedure di assunzione, all'esito degli atti concorsuali, si sono dipanate attraverso diverse fasi finalizzate alla copertura totale dei posti banditi, obiettivo non sempre raggiunto soprattutto nei distretti di corte d'appello dell'Italia del Nord, stante il basso numero dei partecipanti. Alla luce di ciò si specifica che, dopo la prima fase di assunzione dei vincitori, l'amministrazione si è sempre determinata a dare corso a procedure di scorrimento degli idonei residui, operando dapprima nei distretti di corte d'appello con graduatorie capienti e, a seguire, a supporto di quei distretti di corte d'appello privi di candidati idonei, creando graduatorie uniche sulla base del punteggio. In data 6 agosto 2021, con bando delle commissioni Ripam (ente competente per il reclutamento del personale della pubblica amministrazione), è stato indetto un concorso pubblico per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di 8.171 unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale 3, fascia economica F1, con il profilo di addetto all'ufficio per il processo, da inquadrare nel personale del Ministero della giustizia. La procedura si è conclusa con la pubblicazione delle graduatorie di merito e dei vincoli il 14 gennaio 2022. In seguito alla pubblicazione delle graduatorie si è proceduto all'assunzione degli 8.161 vincitori con immissione in servizio dal 14 febbraio 2022. Successivamente, l'amministrazione ha costantemente monitorato l'effettiva copertura dei posti previsti nel profilo di addetto all'ufficio per il processo, così determinandosi ad effettuare tre procedure di scorrimento, a partire dal mese di aprile dell'anno 2022, assegnando 552 unità nella prima procedura, che ha riguardato i distretti di corte d'appello con graduatorie capienti. La seconda procedura è stata effettuata in virtù di quanto previsto dall'articolo 33, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge del 1° marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni dalla legge del 27 aprile 2022, n. 34, con graduatoria unificata agli idonei dei distretti di corte d'appello capienti che, per posizione in graduatoria, non potevano vedersi assegnata la sede a favore dei distretti di corte d'appello le cui graduatorie erano state ampiamente esaurite per scarso numero dei candidati vincitori, per 713 unità. La terza procedura ha riguardato nuovamente i distretti di Corte d'appello con graduatorie ancora capienti, per 462 unità. Considerate le rinunce e le mancate prese di possesso, a fronte di 8.171 posti banditi, sono state assunte 8.157 unità. Gli addetti all'ufficio per il processo, in servizio alla data del 30 giugno 2023, al netto delle dimissioni registrate, risultavano complessivamente 6.113. Vi erano poi 222 idonei non assegnatari di sede nella graduatoria dei distretti di corte d'appello di Bari, Cagliari, Campobasso, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Lecce, Messina, Palermo e Perugia. Questo Dicastero, nelle successive fasi di scorrimento, ha operato seguendo due criteri: il primo, qualitativo, relativamente all'individuazione degli uffici giudiziari da coinvolgere negli scorrimenti, successivamente individuati in uffici giudiziari; il secondo, quantitativo, al fine di determinare il numero delle risorse da assegnare. Nello specifico, le procedure di scorrimento disposte nei mesi di luglio e di agosto dell'anno 2023 hanno portato all'assunzione di 132 unità, con presa di servizio entro il mese di settembre. In ragione della necessità di dare, mediante un nuovo bando concorsuale, piena attuazione alle disposizioni normative che hanno previsto, per il profilo di addetto all'ufficio per il processo, il reclutamento di un contingente massimo di 16.500 unità, l'amministrazione sta esaminando, su tutto il territorio nazionale, le reali esigenze degli uffici giudiziari, anche a fronte delle carenze del personale amministrativo, al fine di definire quali distretti di corte d'appello dovranno essere interessati da un nuovo concorso. È opportuno rammentare ulteriormente che quest'attività di reclutamento affianca, ma non sostituisce, l'ordinaria pianificazione assunzionale. I fondi europei non vanno a finanziare un intervento diretto a colmare le strutturali vacanze del personale, ma si pongono in strettissima e ineludibile relazione con gli specifici obiettivi sopraindicati. Difatti, come più volte ribadito in varie circolari di questo Dicastero, la massiccia immissione di siffatte risorse umane presenta evidenti caratteri di eccezionalità e temporaneità. Questo intervento si fonda dunque su esigenze straordinarie ed è finanziato integralmente con risorse comunitarie, comunitarie, promuovendo i passi entro un segmento temporale ben delineato e non prorogabile. Soltanto previa interlocuzione con la Commissione europea, già avviata da questo Governo, si potrà eventualmente procedere alla stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato. In ogni caso, al termine del contratto di lavoro, l'articolo 3 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, prevede che, al fine di valorizzare l'esperienza professionale maturata nei rapporti di lavoro a tempo determinato, di cui ai commi 4 e 5, lettera *b)*, le amministrazioni di cui al comma 1 prevedano, nei bandi di concorso per il reclutamento di personale a tempo determinato, una riserva di posti in misura non superiore al 40 per cento, destinata al predetto personale che, alla data di pubblicazione del bando, abbia svolto il servizio per almeno trentasei mesi. Inoltre, ulteriori benefici conseguenti al periodo di lavoro presso l'ufficio per il processo sono previsti dall'articolo 11, comma 4, del decreto-legge n. 80 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 113 del 2021, il quale prevede che il servizio prestato con merito e debitamente testato al termine del rapporto di lavoro a tempo determinato, qualora la prestazione lavorativa sia stata svolta per l'intero periodo sempre presso la sede di prima assegnazione, equivalga a un anno di tirocinio professionale per l'accesso alle professioni di avvocato e di notaio, equivalga a un anno di frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali, fermo il superamento delle verifiche intermedie delle prove finali di esame, e costituisca titolo di preferenza per l'accesso alla magistratura onoraria. Oltretutto, il comma 5 dello stesso articolo prevede che l'amministrazione giudiziaria, nelle successive procedure di selezione per il personale a tempo determinato, possa prevedere l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo in favore dei candidati in possesso dell'attestazione di cui al comma 4 ovvero, alternativamente, nei soli concorsi pubblici per le qualifiche della terza professionale, possa prevedere una riserva in favore del personale assunto ai sensi del precedente articolo, in misura non superiore al 50 per cento. Con riferimento agli ulteriori profili trattati nell'atto di sindacato ispettivo, va ricordato che il il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità di questo Dicastero ha segnalato che la figura di dirigente penitenziario è stata istituita, in attuazione della legge delega n. 154 del 2005, col decreto legislativo n. 63 del 2006 e, in forza dell'articolo 3, comma 1-*ter* del decreto legislativo n. 165 del 2001, i dirigenti penitenziari rientrano tra il personale non contrattualizzato di diritto pubblico. Con il DPCM del 15 giugno 2015 n. 84 l'area dell'esecuzione penale esterna è stata trasferita dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità. Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2017 la gestione della dirigenza penitenziaria di esecuzione penale esterna è interamente rimessa al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità. Il successivo decreto legislativo del 29 maggio 2017 n. 95, relativo al riordino delle Forze di polizia, ha stabilito, all'articolo 48, comma 2, che il personale della carriera dirigenziale penitenziaria, fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento degli accordi sindacali prevista dall'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 15 febbraio 2006 n. 63, si applicano gli stessi istituti giuridici ed economici previsti dalla legislazione vigente per il personale della Polizia di Stato appartenente al ruolo di dirigente. La norma assimila quindi lo *status* del personale della dirigenza penitenziaria al personale della Polizia di Stato, non essendo stata ancora istituita l'area negoziale di cui al citato articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 15 febbraio 2006 n. 63. giustizia del 15 febbraio 2019, in attuazione dell'articolo 1, comma 311, della legge del 30 dicembre 2018, n. 145, sette istituti penali per minorenni sono stati classificati quali uffici di livello dirigenziale non generale, inserendo la figura del dirigente penitenziario d'istituto penale per minorenni. In breve tempo, tutti gli istituti penitenziari per minorenni di livello dirigenziale saranno dotati di un dirigente penitenziario titolare. Per ciò che riguarda invece gli istituti penali per minorenni che non sono classificati come sedi dirigenziali, si rappresenta che alla loro direzione è preposto, previo interpello, personale inquadrato nel profilo professionale di direttore Area 3-F4 o, in subordine, nel profilo professionale della professionalità pedagogica Area 3. Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha rimarcato che la contrattazione non può prescindere dalla necessità di uno stanziamento in bilancio di risorse adeguate a coprire tutte le esigenze e le peculiarità di tali categorie, anche in relazione al delicato mandato istituzionale di pertinenza. Ai fini dell'apertura del tavolo contrattuale, si dovrà procedere alla quantificazione a regime delle risorse relative a tutte le componenti del trattamento economico da ritenersi aggiuntive all'attuale spesa concernente le spettanze fisse e continuative con risposta al personale dirigenziale penitenziario, equiparato al primo dirigente della Polizia di Stato, nonché al finanziamento degli importi relativi al periodo di vacanza contrattuale, a partire dall'istituzione della carriera dirigenziale penitenziaria, eventualmente anche a titolo di *una tantum*. L'impegno del Governo è volto a trovare le risorse economiche a questo fine necessarie.

che dichiararmi molto deluso dalla risposta, che mi pare sia stato un grande esempio di burocratese, con una lunga sequenza e un elenco di norme che hanno eluso però completamente i nodi e le questioni politiche che speravamo venissero affrontati, riguardanti una valutazione da parte del Governo sull'ufficio del processo, sulla funzionalità e sull'efficacia di questo strumento che, com'è stato ricordato, è stato introdotto nell'ordinamento dal ministro Orlando nel 2014, ma che in realtà

per un tempo determinato. Sappiamo infatti, com'è stato ricordato, che le risorse del PNRR sono funzionali a un progetto a tempo determinato, quindi non possono essere utilizzate per le assunzioni a tempo indeterminato e questa è una parte del problema. A noi però sarebbe piaciuto capire cosa pensa il Governo dell'ufficio del processo, perché, da quello che risulta a noi - ed è un po' l'auspicio che avevamo, quando anche il Governo Draghi ha deciso di destinare una

Io cito le parole dell'ex primo presidente della Corte di cassazione Pietro Curzio, che ha detto che mediamente gli addetti all'ufficio del processo sono assai più giovani della media del personale della Corte e hanno dimostrato doti che possono rivelarsi molto utili: una grande duttilità di servizio, una forte propensione all'utilizzo degli strumenti tecnologici e una decisa capacità di sfruttare i margini delle attività di cancelleria in chiave di più efficace supporto ai magistrati. tanto vero che nelle prime indagini statistiche che qualcuno ha tentato di fare al Politecnico di Milano sugli uffici di Milano risulta - questo è un dato particolare, ma è stato pubblicato dai giornali pochi mesi fa - che grazie agli addetti all'ufficio del processo a Milano

A me sarebbe piaciuto avere conferma di una valutazione in corso da parte del Ministero sull'efficacia degli addetti all'ufficio del processo, perché questa è la premessa che consideriamo necessaria per arrivare alla conclusione (che anche in questo caso purtroppo è mancata) sulla volontà politica di questo Governo: c'è una volontà politica di questo Governo, al di là dei problemi di natura finanziaria, del fatto che al momento le risorse europee sono limitate e destinate a un'assunzione a tempo determinato? Al di là di questi problemi di natura tecnica, c'è la volontà politica del Governo di prendere atto dell'efficacia dell'ufficio del processo e quindi di garantire la stabilizzazione non dico di tutti, ma di una parte degli addetti all'ufficio del processo? Questo è ciò che a noi interessa e che a noi preme, su cui purtroppo non abbiamo sentito una presa di posizione chiara, nonostante qualche mese fa

penso che tutti quanti (soprattutto noi operatori della giustizia, ma penso tutti i cittadini italiani) abbiamo a cuore l'efficienza della giustizia, che è uno dei principali problemi di questo Paese: sappiamo che condiziona anche l'erogazione del PNRR, ma l'efficienza della giustizia è uno dei principali problemi che riguarda i cittadini italiani. L'ufficio del processo è uno strumento che sta funzionando, pertanto vogliamo sapere se il Governo ha la volontà politica di lavorare in quella direzione per stabilizzare almeno una parte degli addetti che sono stati assunti. La risposta non è arrivata, però noi continueremo a incalzare, perché secondo noi questo è uno strumento indispensabile.

Signor Presidente, onorevoli senatori, la riforma della geografia giudiziaria prevista con la legge delega n. 148 del 2011 ha inteso razionalizzare la dislocazione territoriale degli uffici giudiziari di primo grado, garantendo la permanenza dei tribunali nei Comuni capoluogo di Provincia e assicurando la permanenza di almeno tre tribunali e delle relative procure della Repubblica di ogni distretto di corte d'appello. L'auspicato obiettivo era all'evidenza di *spending review,* riducendo il numero degli uffici giudiziari, con l'allocazione delle risorse disponibili in funzione dei carichi di lavoro. Si deve ritenere che la riforma della geografia giudiziaria non abbia dato gli esiti sperati, pertanto stiamo affrontando siffatta problematica al fine di trovare le soluzioni più idonee. Di recente, sono stati formati dei gruppi di lavoro per verificare la possibilità di conciliare l'efficienza del sistema giudiziario con la doverosa risposta di giustizia di prossimità che lo Stato deve garantire, soprattutto nelle sedi più disagiate. In tale direzione, questo Governo ha già prorogato alla data del 1° gennaio 2025 il rinvio della soppressione dei tribunali di Abruzzo è all'esame la possibile riapertura di uffici giudiziari già soppressi, anche con l'eventuale rimodulazione delle relative competenze territoriali. La priorità del nostro intervento ha anche imposto l'inserimento di un disegno di legge già nel collegato alla legge di bilancio 2023 e quindi nel Documento di economia e finanza licenziato dal Consiglio dei ministri. Per quanto specificamente attiene al distretto di corte di appello dell'Aquila, va ricordato che la riforma della geografia giudiziaria ha in particolare determinato l'accorpamento dei tribunali di Vasto e di Lanciano al tribunale di Chieti, che ha raggiunto i seguenti livelli: 388.280 abitanti, un territorio di 2.588 chilometri quadrati e un indice delle sopravvenienze pari annui. Ha determinato inoltre l'accorpamento dei tribunali di Avezzano e di Sulmona al tribunale dell'Aquila, che ha così raggiunto i seguenti livelli: 297.418 abitanti, un territorio di 5.034 e un indice delle sopravvenienze pari a 15.796 procedimenti annui. Al riguardo, occorre rilevare che risultano presentate diverse iniziative legislative in materia e che, in particolare, presso la 2a Commissione (giustizia) del Senato è in corso l'esame congiunto in sede referente di ben dieci disegni di legge riguardanti una nuova riforma della geografia giudiziaria, essenzialmente volti a ripristinare i presidi in precedenza soppressi e a costituirne di nuovi, di cui sette di iniziativa legislativa regionale. In tale contesto, la Commissione giustizia del Senato, nel corso della seduta del 7 giugno 2023, ha convenuto di costituire un comitato ristretto, incaricato di redigere un testo unificato delle proposte in esame. Dev'essere poi sottolineato che la scopertura media nazionale del personale amministrativo si attesta al 25,74 per cento in relazione alla pianta organica di cui al DPCM del 22 aprile 2022, n. 54. Quanto alle specifiche iniziative poste in essere per far fronte a tale scopertura, corre l'obbligo di evidenziare l'imponente attività di reclutamento che questo Dicastero ha avviato a livello nazionale sin dall'anno 2020. In particolare, siffatto impegno ha consentito l'assunzione di 8.663 risorse umane nell'intero territorio nazionale. Trattasi peraltro di una quantificazione che può definirsi per difetto, in quanto non tiene conto delle assunzioni concernenti gli addetti all'ufficio per il processo e il personale a supporto dell'ufficio per il processo. Di conseguenza, alle citate 8.663 assunzioni dovrebbero essere in realtà aggiunte anche le 12.191 unità relative ai profili di addetto all'ufficio per il processo e di personale a supporto dell'ufficio per il processo, giungendo così a un totale di 20.854 assunzioni. Il distretto di corte d'appello dell'Aquila prevede una pianta organica di 1.056 unità, rispetto alla quale sono coperti 899 posti, con una percentuale di scopertura media del 14,87 (quindi inferiore rispetto alla media nazionale). Tale distretto comprende allo stato 43 uffici giudiziari, ripartiti tra la città capoluogo (sede di dieci uffici) e otto circondari; tuttavia, per effetto del decreto legislativo n. 155 del 2012, è prevista la soppressione, alla data dell'1° gennaio 2025, dei tribunali e delle procure della Repubblica di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto e il loro accorpamento agli uffici dell'Aquila (Avezzano e Sulmona) e Chieti (Lanciano e Vasto). del 19 maggio 2015 le piante organiche degli uffici giudiziari di tutto il territorio nazionale sono state riorganizzate: a fronte dell'incremento dei posti negli organici degli uffici giudiziari accorpanti e nel rispetto dell'invarianza della dotazione organica complessiva nazionale, sono state annullate le piante organiche degli uffici giudiziari

Quanto agli uffici giudiziari accorpanti, i relativi organici sono stati incrementati tenendo già conto della situazione che si determinerà quando il personale degli uffici giudiziari in soppressione sarà assegnato agli stessi.

l'accertamento dell'illegittimità del silenzio del Ministero della giustizia in relazione all'invito a procedere alla copertura di tutti i posti del personale amministrativo vacanti nel tribunale di Avezzano. dell'Abruzzo ha ritenuto fondato nel merito il ricorso e dichiarato l'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero della giustizia sull'istanza del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Avezzano del 29 agosto 2022, ordinando di provvedere sulla stessa entro trenta giorni dalla notifica della sentenza. In proposito bisogna sottolineare che la citata decisione del giudice amministrativo ha come riferimento il tribunale di Avezzano e il mancato pieno riscontro dell'amministrazione «(...) all'istanza del Consiglio, corredata da dati che dimostrano l'inefficienza del Tribunale di Avezzano imputabile alla carenza di personale dipendente dell'area amministrativa e chiaramente intesa a sollecitare l'adozione degli atti necessari a garantirne la funzionalità (...)», non ponendo alcun diretto obbligo di ricostituzione della pianta organica del presidio giudicante o di copertura della stessa, come determinata precedentemente alla relativa soppressione, atteso che «(...) la verifica dell'adeguatezza delle risorse assegnate agli Uffici Amministrativi costituisce esercizio di attività ampiamente discrezionale

convertito con modificazioni dalla legge n. 74 del 2023, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, non prevede l'obbligo, ma solo la possibilità per l'amministrazione di valutare l'adozione degli interventi ritenuti opportuni in materia di adeguamento dell'organico del personale amministrativo dei tribunali soppressi delle circoscrizioni dell'Aquila e di Chieti, in funzione del conseguimento degli obiettivi posti per la giustizia nell'ambito del Piano In ogni caso, va segnalato che nel distretto di corte d'appello dell'Aquila, a partire dall'anno 2020, sono state effettuate 312 assunzioni, cui ne vanno aggiunte altre 309 con contratto a tempo determinato di addetti all'ufficio per il processo e di personale a supporto dell'ufficio per il processo. Altresì, con provvedimento del 10 novembre 2022 è stato dato l'avvio alla procedura di stabilizzazione del personale in servizio nella qualifica di operatore giudiziario, che ha visto partecipare nel distretto di corte d'appello dell'Aquila 39 unità di personale con presa di possesso nel mese di gennaio 2023 e un'ulteriore unità avrà la possibilità di essere stabilizzata alla prevista scadenza contrattuale. Si rileva poi che nel distretto di corte d'appello dell'Aquila, con provvedimento del direttore generale del 20 giugno 2023, sono stati resi disponibili ulteriori otto posti di cancelliere esperto dal concorso a 2.700 unità per scorrimento della graduatoria. Tra il 10 e il 20 luglio 2023 i candidati all'assunzione sono stati invitati a scegliere la sede di lavoro tra quelle messe a disposizione dall'amministrazione. All'esito della procedura di scelta, con avviso del 2 agosto 2023, sono stati resi noti i nominativi degli idonei che avrebbero dovuto sottoscrivere il contratto individuale di lavoro in data 5 settembre 2023 nei seguenti uffici giudiziari: tribunale di Vasto, un'unità; tribunale dell'Aquila, due unità; tribunale di Avezzano, un'unità; procura della Repubblica presso il tribunale dell'Aquila, un'unità; tribunale di Pescara, un'unità; tribunale di Chieti, un'unità, e procura della Repubblica presso il tribunale di Pescara, un'unità. Sebbene il posto reso disponibile nel tribunale di Avezzano sia stato oggetto di scelta da parte di un idoneo presente in graduatoria, alla data prevista per l'immissione in possesso non è stato coperto dall'avente diritto; di contro, al tribunale di Vasto si è proceduto alla prevista assunzione di una risorsa umana. Per quanto concerne le posizioni dirigenziali, si segnala che, su nove posti disponibili, quattro sono coperti con incarico di titolarità e uno con incarico di reggenza. Tutte le posizioni vacanti sono state pubblicate con interpello del 10 maggio 2023. In data 26 luglio 2023 è stato pubblicato l'interpello ordinario nazionale per 9.739 posti vacanti rivolto al personale dell'organizzazione giudiziaria, ai sensi dell'articolo 4 dell'accordo sindacale del 15 luglio 2020. Per la Regione Abruzzo nel suo complesso sono stati resi disponibili 279 posti. Nell'introduzione al bando di interpello si legge: «(...) in relazione agli Uffici Giudiziari sopprimendi della Regione Abruzzo vengono pubblicati posti negli Uffici accorpanti con assegnazione agli Uffici accorpati fino alla data di effettiva chiusura dei medesimi (...)». Si rimarca a questo punto che dal Piano triennale dei fabbisogni 2023-2025 emerge chiaramente la volontà di questo Dicastero di sopperire quanto più possibile alle carenze di personale amministrativo. Le attività di reclutamento previste nell'arco temporale che va dal 2023 al 2025 concernono complessivamente 1.051 unità

non dirigenziale, per le quali l'autorizzazione a bandire e ad assumere, in aggiunta alle facoltà assunzionali, è prevista da varie fonti normative, divise in 1.967 funzionari e 1.724 assistenti. Si evidenzia infine che, allo scopo di fronteggiare le ulteriori criticità che nel frattempo dovessero sopravvenire, determinate dal pensionamento di unità di personale ovvero da altre situazioni soggettive di carattere temporaneo (maternità, malattia eccetera), l'organico del personale amministrativo degli uffici giudiziari in difficoltà potrà essere implementato facendo ricorso all'istituto della mobilità temporanea del personale, previsto dall'articolo 20 dell'accordo sottoscritto in data 15 luglio 2020, come modificato dall'*addendum* sottoscritto il 22 marzo 2023.

Questa risposta, un po' come la precedente, è il massimo del burocratismo e dice, fra le altre cose, che ci si occuperà di far fronte all'esigenza di fare la revisione alla riforma della geografia giudiziaria, si è aperta la discussione in Commissione, ci sono molte proposte di legge e si è creato un sottogruppo di lavoro, una sottocommissione di cui fa parte il senatore Verini. Va bene, ma naturalmente ci aspettiamo che ci sia una verifica, dopo oltre dieci anni, di che cosa è accaduto laddove i tribunali sono stati chiusi e dell'esito rispetto all'obiettivo che ci si era dati. Si fa il punto

Nello specifico, però, stiamo parlando di una situazione del tutto particolare, non assimilabile alle altre, perché in Italia ci sono territori in cui i tribunali sono rimasti aperti e altri in cui sono stati chiusi. Solo in questo caso, invece, è stato stabilito sulla carta che alcuni tribunali dovessero chiudere e per dieci anni, con dieci anni di proroghe, invece sono rimasti aperti. di quattro tribunali, Avezzano, Sulmona, Vasto e Lanciano, che naturalmente hanno continuato a lavorare esattamente come lavoravano prima. Tutte le risposte relative all'assunzione di personale e all'ufficio del processo, sulle quali possiamo discutere, non riguardano la mia interrogazione, che verte invece su che cosa sta accadendo in questi tribunali in relazione al personale. punto la risposta, nel massimo del burocratese, è agghiacciante: questi tribunali sono stati chiusi sulla carta, quindi non hanno pianta organica e li si considera chiusi, solo temporaneamente rimasti aperti. La logica vorrebbe che li considerassimo aperti finché una decisione definitiva, che io spero non ci sia mai, non li chiuda. Mi viene in mente uno *sketch* straordinario tra Troisi, Arbore e Frassica, in cui Arbore aveva scritto sulla carta che Troisi non era Troisi, ma era un altro attore e cercava di convincerlo che lui era quello e che doveva essere contento. Noi quindi dobbiamo provare a convincere questi tribunali che continuano a lavorare che in realtà sono chiusi,

La media della copertura nel distretto dell'Aquila è del 14 per cento. In questa interrogazione c'è scritto quindi che la scopertura rispetto alla pianta organica del 2009 (che adesso non si può più nemmeno chiamare pianta organica, perché non hanno diritto ad averla),

e naturalmente il Ministero risponderà: il TAR si faccia i fatti suoi, noi la pensiamo così. Di fatto, stiamo garantendo un cattivo servizio della giustizia. Mentre ci occupiamo di risolvere definitivamente questo problema, decidendo se questi tribunali devono restare

ha la sua pianta organica e viene considerato come tale. Viene considerato senza pianta organica solo nel momento in cui chiude. È questo che direbbe chiunque con un po' di buon senso, guardando la realtà prima delle carte.

in località Casalborsetti è di proprietà del Comune di Ravenna e confina con un villaggio turistico privato. L'area suddetta è ubicata all'interno del parco regionale del Delta del Po tra le zone classificate come aree agricole da privilegiare per il ripristino naturalistico, per le quali sono previsti il mantenimento e la conservazione di rari esempi di successione naturale di *habitat* costieri, dunali e retrodunali. Segnatamente, si tratta di area rientrante nel perimetro della zona speciale di conservazione, zona di protezione speciale IT407005, in Pineta di Casalborsetti, Pineta Staggioni Duna di Porto Corsini. Risultano inclusi tre *habitat* di interesse comunitario con presenza di dune, nonché di vegetazione con pini marittimi e pioppi bianchi. Si evidenzia al riguardo che l'area non è visibile dalla pubblica via. L'accesso alle zone in cui insistono i capanni e in quelle limitrofe è possibile tramite uno stradello sterrato che costeggia il fiume Lamone ed è poi necessario proseguire a piedi a nord del villaggio. Competente alla vigilanza sull'area è la stazione dei Carabinieri forestali di Ravenna. Su tutta la fascia boscata ubicata lungo la costa, immediatamente a est di quella all'esame, è competente il Nucleo tutela biodiversità di Casalborsetti, a cui spetta il controllo e il monitoraggio della riserva naturale Pineta di Ravenna. A seguito di segnalazione del dirigente del Servizio tutela ambientale del comune di Ravenna, lo scorso 3 marzo 2023, la citata stazione di Ravenna competente per territorio è intervenuta per accertamenti, riscontrando l'esecuzione di lavori di movimentazione terreno e taglio di vegetazione in assenza di autorizzazione in area naturale protetta, sottoposta a vincolo idrogeologico e paesaggistico. L'intervento ha comportato la completa eliminazione della vegetazione arborea, arbustiva ed erbacea per una fascia di larghezza variabile dai 15 ai 30 metri. Il terreno di risulta derivante dalle operazioni di decorticazione è stato addossato alla vegetazione limitrofa non interessata dall'intervento. Per quanto riguarda la componente arborea, è stato accertato il taglio di esemplari di pino domestico adulto e parte di una giovane fustata di pioppo bianco. L'area di 7.700 metri quadrati, unitamente ad una catasta di circa 45 metri cubi di legname depezzato, veniva immediatamente sottoposta a sequestro. Le ipotesi di reato sono per deterioramento di *habitat* all'interno di un sito protetto, ai sensi dell'articolo 733-*bis* del codice penale, e per esecuzione di lavoro in assenza di permesso di costruire in area sottoposta a vincolo paesaggistico n. 380 del 2001, articolo 44, comma 1, lettera *c)*. Nei giorni successivi, il sequestro è stato convalidato dall'autorità giudiziaria. Il reparto operante ha tempestivamente avviato le attività le attività di indagine finalizzate ad individuare le responsabilità dell'azione illecita. Delle notizie acquisite a seguito degli accertamenti svolti, che sono attualmente soggette a segreto istruttorio, ai sensi dell'articolo 229 del codice di procedura penale, veniva data comunicazione all'autorità giudiziaria. La notizia dell'accaduto ha avuto ampio risalto da parte degli organi di informazione locale. Il sindaco di Ravenna ha dichiarato pubblicamente di avere già provveduto a richiedere alla procura della Repubblica l'accesso all'area per effettuare un sopralluogo finalizzato alla progettazione della ripiantumazione, non appena le condizioni stagionali lo permetteranno, presumibilmente a partire già dal prossimo autunno. Le possibili azioni di ripristino dell'area dovranno essere definite a valle delle conclusioni di tali accertamenti. In ogni caso, i relativi costi dovranno essere posti in capo all'esecutore degli interventi attuati in presunta difformità dalle previsioni di legge. Ferme restando le conclusioni circa le responsabilità degli esecutori del danno, il Ministero conferma la disponibilità nel seguire gli sviluppi della vicenda e, parimenti, a rendersi parte attiva durante le fasi di ripristino delle condizioni naturali nell'area

di favorire gli *habitat* naturali e le biodiversità del territorio, tutelandole anche con normative specifiche. Dobbiamo trovare il modo di investire continuamente nella tutela del territorio ed incrementare gli spazi di biodiversità. La pineta è amata dai ravennati, ma è apprezzata dai turisti di tutta Italia e di tutta Europa, quindi ogni centesimo investito per tutelare e salvaguardare quel territorio sicuramente avrà una ricaduta su tutta la comunità, anche internazionale. Come monito

le attività previste sono state in massima parte attuate e concluse o sono in corso di realizzazione. In particolare, su sedici progetti, dieci sono conclusi, cinque sono in corso e uno è in valutazione. Per completezza, dati i limiti di tempo, consegno agli atti, a disposizione dell'interrogante e dei colleghi interessati, una tabella dettagliata. Quanto al quesito sulla programmazione dei progetti dedicati alle persone LGBT nel Piano nazionale di inclusione e lotta alla povertà 2021-2027, si informa che l'UNAR ha partecipato agli incontri con gli altri soggetti istituzionali coinvolti sul tema degli adempimenti per il soddisfacimento delle cosiddette condizioni condizioni abilitanti, tra le quali rientra anche l'adozione della strategia nazionale LGBT+. L'UNAR inoltre ha collaborato con il nucleo di valutazione e analisi per la programmazione delle politiche di coesione e di sviluppo territoriale, nella definizione degli indicatori comuni di *output* per misurare i risultati degli interventi. Per identificare le tipologie di azione da proporre nella nuova programmazione, nel marzo 2022 sono state trasmesse, all'autorità di gestione del programma nazionale inclusione e lotta alla povertà, le schede di rilevazione delle azioni da attuare per i *target* vulnerabili di competenza, tra cui le persone LGBT+. Le azioni si allineano agli obiettivi e alle misure definiti dalla Strategia europea per l'uguaglianza delle persone LGBT+ 2020-2025 e dalla Strategia nazionale 2022-2025. A seguito dell'approvazione del Piano nazionale inclusione e lotta alla povertà 2021-2027 da parte della Commissione europea, il 1o dicembre 2022, nelle prossime settimane l'UNAR procederà alla sottoscrizione della convenzione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il cui piano operativo e progettuale è in corso di definizione. In riferimento al portale nazionale LGBT+ e alla pubblicazione del materiale derivante dalla digitalizzazione degli archivi storici, l'UNAR ha proceduto con un intervento di riprogettazione e realizzazione dell'infrastruttura tecnico-informatica, implementando il portale preesistente e creando una sezione archivio per il materiale storico-documentario. Portale e archivi saranno *online* al termine dell'attività di revisione, riorganizzazione e implementazione dei contenuti redazionali, entro dicembre 2023. Per quanto riguarda i centri contro le discriminazioni LGBT+, in attuazione della normativa vigente, è stato acquisito, nella seduta del 10 maggio 2023, il parere favorevole della Conferenza unificata sullo schema di decreto per il rinnovo delle convenzioni stipulate all'esito dell'avviso del 10 marzo 2021 per la gestione dei centri già esistenti, mediante le risorse stanziate per l'anno 2021. Comunico inoltre che il 23 maggio scorso ho firmato il decreto che ha consentito lo sblocco dei fondi 2020-2021, dando continuità alle progettualità realizzate. L'UNAR ha proceduto alla pubblicazione del decreto e dato avvio alla procedura amministrativa per l'erogazione dei fondi ai beneficiari, tramite la stipula delle nuove convenzioni. Con i nuovi progetti vi sarà anche l'acquisizione di un flusso dati finora mancante, per individuare esigenze concrete e risposte più efficaci possibili per la tutela delle vittime di discriminazione. Si procederà successivamente, all'esito della sperimentazione della seconda annualità, all'utilizzo delle risorse previste per gli anni 2022 e 2023. e 2023. Quanto ai centri finanziati in base all'avviso 2021, con le risorse dell'anno 2020, si rappresenta che, su 46 centri, 42 hanno concluso l'attività, mentre i rimanenti sono in corso. Veniamo alla richiesta di informazioni sulle iniziative svolte in occasione del 17 maggio, Giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia. Per la Giornata internazionale, l'UNAR ha realizzato la campagna di sensibilizzazione, della durata di sei mesi, con il *claim*: "#unosguardoin+", per la libertà di tutte le persone, nella loro unicità, di essere pienamente se stesse. Da menzionare inoltre la campagna promossa dalla Lega Serie A e da UNAR nell'ambito del protocollo d'intesa siglato lo scorso 14 marzo, contro ogni forma di discriminazione nel mondo del calcio. Concludendo, colgo l'occasione per ricordare, in materia di tutela delle libertà e della lotta alle discriminazioni, che il Senato ha votato una mozione unitaria sul contrasto all'omofobia, con il parere favorevole del Governo.

a questa interrogazione, cosa che gli altri Ministri - lo devo riconoscere - non hanno fatto. Il fatto che i fondi destinati ai progetti e ai centri di tutela delle persone LGBT siano stati finalmente sbloccati a maggio scorso - devo dirlo - ha fatto tirare un bel sospiro di sollievo sollievo naturalmente alle persone vittime di violenza, che hanno la possibilità di accedere ai centri, alle associazioni che se ne occupano, ma anche a noi, come MoVimento 5 Stelle in particolare. L'istituzione del fondo, avvenuta nel 2020, sotto il Governo Conte, rappresenta una piccola rivoluzione, di cui siamo estremamente orgogliosi, per diversi motivi. Innanzitutto, rappresenta l'unico gesto concreto che la politica abbia fatto nei confronti delle persone LGBT per anni. Inoltre, l'esistenza stessa di questi centri, Ministra, testimonia due cose. Da una parte, testimonia

c'è la volontà della Repubblica di adempiere a un compito che la Costituzione le assegna, e cioè rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona. Questi centri, quindi, non sono

per questo sono particolarmente orgogliosa. C'è un'altra caratteristica che marca l'istituzione di questi centri e dei fondi così come li abbiamo voluti.

quindi che la prossima assegnazione, quella che riguarderà il 2022, avverrà tramite bando e non tramite rifinanziamento dei vincitori del bando precedente. Lo spirito dell'istituzione di questi fondi consiste, infatti, proprio nel consentire la nascita di altri che siano semplicemente sportelli di assistenza legale, psicologica e sanitaria, o centri presso i quali le persone possono anche essere ospitate. Purtroppo sappiamo che nel nostro Paese capita ancora troppo di frequente che ragazzi e ragazze, anche giovanissimi, vengano disconosciuti e cacciati dalla propria famiglia per il loro orientamento sessuale o identità di genere. Lo spirito dunque è questo e mi auguro che i prossimi fondi vengano erogati attraverso bando, proprio per consentire la nascita di altri centri.

al libro pubblicato da un tal generale, che ha affermato che le persone LGBT non sono normali: il ministro Crosetto è stato lasciato da solo a stigmatizzare la gravità di tali affermazioni antiscientifiche, che vanno contro ogni cognizione fondata scientificamente

anche in quel caso non ricordiamo interventi a tutela da parte sua.

a valle, se vogliamo provare davvero a contrastare la violenza, sia essa contro le donne o violenza e discriminazione contro le persone LGBT, lei sa bene quanto me che l'unico intervento da fare è nelle scuole. La mia proposta è quindi la seguente: impegniamoci tutte e tutti insieme per inserire all'interno delle nostre scuole dei percorsi di educazione sessuale ed emotiva. Soltanto andando alla radice

finestra") sulla nomina di un diplomatico italiano al vertice della delegazione di Tripoli del servizio esterno dell'Unione europea,

nella nostra politica estera, su un Paese strategico come la Libia, che sarebbe veramente preoccupante. Cerchiamo di riassumere brevemente cosa è successo anche per chi ci segue da casa. Un diplomatico italiano partecipa alla selezione per diventare l'ambasciatore dell'Unione europea a Tripoli e vince la selezione. L'esito della selezione gli viene comunicato nel mese di aprile. Che cosa succede, però, dal mese di aprile? Niente. Egli dovrebbe assumere la posizione dal 1° settembre, ma non accade nulla. I giornali, però, raccontano che, tra il 7 e l'8 giugno, il Primo Ministro libico viene a Roma e comunica all'Italia che non darà il gradimento a questo ambasciatore. Questa è una cosa gravissima nel galateo diplomatico. Non si usa. Il mancato gradimento è proprio uno schiaffo in faccia a un Paese. Stranamente, però, quello che accade è che non accade niente, tant'è che il mancato gradimento, annunciato verbalmente, viene messo per iscritto in una nota verbale che va all'Unione europea.

e la sede resta vacante. I giornali italiani scoprono allora la vicenda e la raccontano, parlando appunto di uno schiaffo in faccia a Meloni. Bastano pochi articoli sui giornali italiani e qualcuno, purtroppo, anche sui giornali internazionali perché il Governo libico cambi idea e dia dia il gradimento al nostro diplomatico; ciò a dimostrazione che, se il suo Ministero si fosse mosso, noi ci saremmo evitati uno schiaffo in faccia dalla Libia: tra l'altro per mandarci un francese. E Dio solo sa che, se c'è un Paese che proprio non ha interessi convergenti con noi sulla Libia, quella è la Francia. La vostra inazione è anche dimostrata da un incredibile dichiarazione che lei ha rilasciato al *meeting* di Cernobbio, che leggo perché merita. Ella dice ai giornalisti: «Non c'è alcun candidato italiano. Non bisogna confondere l'Italia con l'Unione europea». Quindi, il Ministro degli affari esteri italiano afferma che non bisogna confondere l'Italia con l'Unione europea. con l'Unione europea. Una questione riguardante i rappresentanti del servizio esterno dell'Unione europea è una questione che non riguarda l'Italia. Quindi, se a Tripoli c'è un italiano o un francese, per lei è la stessa cosa. Io vorrei sapere, innanzitutto, se la storia è vera; è vera; perché non vi siete mossi quando ufficiosamente vi è stato detto che il gradimento non c'era; perché non avete fatto sentire un po' la vostra voce, come si fa tra Governi amici. E noi il Governo libico l'abbiamo molto sostenuto. In secondo luogo, chiedo se è vero che non c'era un candidato italiano. Da *ex* Sottosegretario al Ministero degli affari esteri, infatti, io so che i nostri diplomatici vengono scelti e sostenuti dalla Farnesina: non si alzano la mattina e si iscrivono a una selezione. Da ultimo, signor Ministro, chiedo che cosa sta facendo ora per fare in modo che sia un italiano a ricoprire quel posto, visto che l'Unione europea aveva già allertato un francese. Chi ci va adesso? L'italiano o il francese? Insomma, riesce a rimettere il dentifricio nel tubetto e a sistemare il guaio che ha combinato?

dei rapporti con l'Unione europea. Esiste, infatti, una diplomazia dell'Unione europea che è diversa dalla diplomazia di ogni singolo Stato membro, che svolge anche attività diverse, in nome e per conto dell'Unione europea e non in nome e per conto dello Stato membro. Anzi, i diplomatici che appartengono a quella diplomazia non devono fare l'interesse nazionale, ma devono svolgere l'interesse dell'Unione europea. Un europeista come lei dovrebbe sapere anche questo. L'ambasciatore d'Italia Gianluca Albertini, nominato dal Governo, ha ottenuto immediatamente il gradimento da parte del Governo libico; quindi non c'è alcun atteggiamento negativo nei confronti

di non prendere ordini dal Governo. Quindi l'ambasciatore dell'Unione europea non deve prendere ordini dal Governo italiano e lei questo lo sa molto bene. Ciò è tanto vero che noi siamo stati soddisfatti quando il servizio esterno ha deciso di candidare il consigliere Orlando, che, dopo un iniziale diniego, ha poi ottenuto l'autorizzazione da parte del Governo libico e quindi sarà lui il futuro futuro rappresentante dell'Unione europea presso il Governo di Tripoli. Si è trattato di una tempesta in un bicchier d'acqua, che ha il sapore un po' della polemica politica. Per carità, la polemica è il sale della democrazia, ma le regole sono le regole e le istituzioni sono le istituzioni. Noi rispettiamo l'Unione europea e così abbiamo fatto. Continueremo ad avere buoni rapporti con la Libia e, rispondendo alle successive interrogazioni, dirò anche quello che stiamo facendo per aiutare il popolo libico in questo momento. Ribadisco, il servizio esterno dell'Unione europea è una cosa e la diplomazia della Repubblica italiana è un'altra: non sono due cose che si intrecciano e si mischiano. Anche se il diplomatico è italiano, deve rispondere all'autorità comunitaria ed è al servizio dell'intera Unione europea e non al servizio esclusivo dell'Italia. Gliel'ho dovuto ricordare perché, dopo un po' di tempo che non sta al Ministero, forse se l'era dimenticato.

da lei e dai suoi colleghi del Governo perché faccia gli interessi dell'Italia. *(Applausi)*. Quindi può darsi che io mi sia dimenticato qualcosa, perché sono lontano dalla Farnesina da un paio d'anni, ma lei che ci sta dentro, pur essendo nella Farnesina, non se ne ricorda. Per Per consolarlo e tirarlo su di morale, manderò questa registrazione al commissario Gentiloni. Detto questo, ci sono comunque delle cose che non tornano. Innanzitutto lei non ci ha detto perché la Libia non ha dato il gradimento al nostro ambasciatore, mettendolo addirittura per iscritto. Probabilmente - dicono i giornali - i francesi hanno un Ministero degli esteri un po' più efficace, che pensa invece che sia interesse della Francia che il rappresentante *in loco* sia francese e non italiano, perché altrimenti è un mistero. L'approssimazione e il dilettantismo sulla Libia non li dimostra soltanto questa piccola storia, ma, molto più gravemente, il grave incidente diplomatico che si è verificato tra Libia e Israele, quando il suo Governo ha organizzato in questo Paese, a Roma, un incontro che poi gli israeliani hanno reso noto alla Libia e al mondo intero. Allora io mi chiedo: ma quando lei riceve una delegazione per un incontro così delicato, lei prenota soltanto le automobili e gli alberghi o si preoccupa di fare in modo che la la riunione nella sua interezza sia gestita in modo adeguato? Signor Ministro, lei ha detto che voi siete tornati protagonisti in politica estera. Ma, se io considero queste vicende, e ci aggiungo il famoso piano Mattei, che ancora nessuno ha mai visto - tutti ne parlano, come l'araba fenice, ma non lo si è mai visto - ho dei grandi dubbi che la politica estera di questo Paese ci faccia tornare ad essere protagonisti, in particolare in Libia.

*(FI-BP-PPE)*. Rimaniamo sul tema della Libia, per affrontare una questione assai drammatica. Come credo sia noto a tutti, il ciclone Daniel ha creato delle piogge torrenziali, che hanno interessato in particolare la cirenaica e che hanno portato, soprattutto nella città di Derna, a un'autentica catastrofe (si parla addirittura di 20.000 morti, oltre a distruzioni, feriti, dispersi e danni materiali). È del tutto evidente che questo è dipeso da un fenomeno climatico eccezionale, ma anche, in particolare, dallo stato di alcune dighe, che da tempo non ricevevano della manutenzione e quindi sono crollate e hanno portato al disastro che abbiamo capito essere successo. E questo dipende - come sappiamo bene - soprattutto dall'instabilità politica che interessa quell'area e dalle guerre che si sono succedute. Ricordiamo tra l'altro che Derna era anche una delle capitali dell'Isis in quel contesto. L'Italia ha degli interessi e dei legami storici e

a lei, signor Ministro, quali sono le iniziative immediate e anche di prospettiva che il nostro Governo intende mettere in campo per aiutare e sostenere quelle popolazioni così martoriate. PRESIDENTE.

senatore Scalfarotto, che è così interessato ai problemi della Libia, quando si parla di un disastro abbia abbandonato l'Aula; forse ci seguirà attraverso la televisione, com'è suo costume. La Libia sta attraversando giorni drammatici: il ciclone Daniel si è abbattuto su un Paese già ferito e sofferente e le immagini del disastro sono strazianti. Siamo vicini al popolo libico e alle famiglie delle tante vittime. La perturbazione ha colpito in particolare l'area costiera della Cirenaica. L'inondazione generata dal collasso di due dighe ha devastato la città di Derna, simbolo di questa catastrofe umanitaria. Le stime parlano di decine di migliaia di morti e dispersi, purtroppo in continuo aggiornamento. La nostra ambasciata a Tripoli, il consolato generale a Bengasi e la Protezione civile verificano costantemente la situazione dei connazionali presenti nella regione. Parte di una famiglia italo-libica risulta ancora dispersa: i due figli maggiori sono stati appena rintracciati, sono vivi e a casa dei nonni. Per i genitori e la figlia più piccola le ricerche proseguono senza sosta. Restiamo in contatto con i parenti. Le operazioni di soccorso procedono in condizioni difficili, le autorità libiche hanno chiesto subito aiuto alla comunità internazionale e all'Italia in particolare. Insieme al Presidente del Consiglio abbiamo assicurato aiuti e vicinanza. Ho subito dato istruzione di rispondere con massima sollecitudine alla richiesta di sostegno. Abbiamo istituito un coordinamento tra Ministero degli affari esteri, Protezione civile, Comando operativo vertice interforze e Vigili del fuoco. Martedì una squadra coordinata dalla Protezione civile ha effettuato a Derna una prima ricognizione per stabilire i collegamenti operativi con le autorità locali e definire gli aspetti tecnici della risposta italiana. Ieri due nostri voli hanno trasportato squadre specializzate, attrezzature di supporto e materiale di prima necessità; un terzo volo è stato effettuato questa mattina. La nave San Giorgio della Marina militare è già al largo di Derna e assicurerà le funzioni logistiche di comando e controllo, oltre che di supporto sanitario al dispositivo nazionale. La nave San Marco è in navigazione; a bordo sono stati caricati elicotteri per attività di ricerca e soccorso, mezzi di movimento terra, cento tende da campo, mille brandine con sacchi a pelo e ulteriori squadre specializzate. Abbiamo offerto personale, beni e materiali anche nel quadro delle iniziative coordinate a livello europeo. Il Governo ha disposto un primo contributo di 350.000 euro sui fondi immediatamente disponibili nell'ambito della risposta umanitaria delle Nazioni Unite. Alla luce della gravità della situazione intendiamo erogare ulteriori fondi. Continueremo a seguire la situazione sul terreno e in stretto contatto con le autorità locali, le agenzie internazionali e gli altri *partner*. Nelle prossime ore è prevista una missione anche del capo dipartimento della protezione civile Fabrizio Curcio nelle aree colpite. Vogliamo contribuire concretamente ad aiutare un Paese *partner* e un popolo amico.

del nostro Paese nei confronti delle popolazioni colpite, con le quali - come dicevo prima - siamo legati da vincoli di amicizia storici ed anche economici. Tante volte abbiamo detto che la stabilità e la prosperità dell'Europa dipendono soltanto dalla prosperità e dalla stabilità del lato Sud del Mediterraneo. Questa, quindi, può essere un'occasione per riannodare dei fili che sono storici, che ci appartengono, per aiutare quelle popolazioni e per favorire anche quella politica di pace che tante volte la nostra diplomazia ha cercato di supportare in quelle aree, anche se fino ad oggi non ci siamo riusciti, e anche riusciti, e anche per cercare di contenere l'espansionismo russo e dei mercenari della Wagner in quel settore così strategico per i nostri interessi economici. L'auspicio è che, di fronte a una situazione così drammatica, a una catastrofe umanitaria che è anche legata a quella climatica, possano trovare

Premesso che: come riportato da numerosi organi di stampa, il finanziamento pubblico al Servizio sanitario nazionale è stato decurtato, decurtato, negli anni 2010-2019 in valore assoluto, di oltre 37 miliardi di euro, dei quali circa 25 miliardi nel 2010-2015 per tagli conseguenti a varie leggi di bilancio ed oltre 12 miliardi nel 2015-2019, quando alla salute sono state destinate meno risorse di quelle programmate per esigenze di finanza pubblica; in particolare, il finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* ha addirittura, negli anni dal 2012 al 2019, visto decrementi annui

dal 2019 al 2022, hanno previsto un aumento del fabbisogno del Servizio sanitario nazionale, ma possono essere considerati "bilanci di guerra" dal momento che si sono dovuti fronteggiare i costi dovuti dall'emergenza epidemiologica

effettivi; nonostante la grave situazione pregressa descritta e nonostante le oggettive difficoltà economiche, dovute alla crisi energetica, alla guerra russo-ucraina, all'aumento di costi delle materie prime, questo Governo ha aumentato le risorse destinate si ritiene, tuttavia, necessario realizzare ulteriori innovativi e maggiori interventi, per raggiungere un valore di finanziamento del FSN rispondente all'effettiva domanda di salute del nostro Paese,

quello del giusto livello di finanziamento del nostro Sistema sanitario nazionale, tema tuttavia che è stato e viene ancora utilizzato da taluni in maniera erronea e fuorviante. In termini di valore assoluto, il finanziamento del fondo sanitario nazionale *standard* ha vissuto stagioni non troppo lontane di valori negativi in cui il fondo nazionale è stato effettivamente tagliato o definanziato. Come giustamente sottolineato dagli interroganti, il fondo ha visto incrementi annui in valore percentuale negativo dello 0,89 nel 2013, del meno 0,19 nel 2015, appena dello 0,73 nel 2018 e dello 0,94 nel 2019. Di contro la prima legge di bilancio del Governo nel 2023 ha previsto un incremento del fondo sanitario nazionale. Al comma 535 dell'articolo 1 è disposto che il finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* incrementato di 2 miliardi e 150 milioni per l'anno 2023, 2 miliardi e 300 milioni per l'anno 2024, 2 miliardi e 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Inoltre, per l'anno 2023 l'articolo 8 del decreto-legge n. 34 del 2023, convertito dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, ha ulteriormente finanziato per un miliardo e 255 milioni di euro la spesa sanitaria nazionale, in parte per far fronte alla problematica del cosiddetto *payback* dei dispositivi medici - anche questa ereditata dai Governi precedenti - in parte per implementare la tariffa oraria delle prestazioni aggiuntive, anticipare l'indennità nei servizi di emergenza e urgenza al fine di contrastare il fenomeno del ricorso ai cosiddetti medicini gettonisti. In effetti per l'anno corrente si è registrato, nonostante le oggettive difficoltà economiche, un incremento inedito di oltre 3 miliardi di euro dal livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale pari a circa il 3 per cento, inferiore solo a quello registratosi nell'anno 2020 a causa dello straordinario sforzo finanziario richiesto per fronteggiare i maggiori costi legati all'emergenza Covid. Devo inoltre ricordare che, nell'ambito del PNRR per l'attuazione delle Missione 6 salute, è previsto un finanziamento pari a 15,63 miliardi di euro ai quali si sommano 1,71 miliardi del fondo React-EU e 2,89 miliardi di euro del fondo complementare. L'investimento prevede l'acquisto di nuove e grandi apparecchiature ad alto contenuto tecnologico, digitalizzazione di ospedali, istituzione di case di comunità, ospedali di comunità e centrali operative e territoriali. Sono tutte azioni in continuità e coerenti con gli investimenti previsti nel Patto della salute. quindi di risorse nel complesso importanti, che riteniamo però ancora necessario implementare per garantire un livello di qualità elevata del Servizio sanitario nazionale e di risposta ottimale ai bisogni di salute della collettività. Per questi motivi è in corso una serrata e proficua interlocuzione nel Governo, soprattutto con il Ministero dell'economia e delle finanze, affinché la prossima legge di bilancio destini ulteriori e importanti risorse al Sistema sanitario nazionale da rivolgere anche al miglioramento del trattamento economico dei professionisti del settore pubblico, che deve essere reso più appetibile, e all'abbattimento delle odiose liste d'attesa. In questo senso ben venga ogni iniziativa parlamentare finalizzata a individuare ulteriori fonti di finanziamento, quale ad esempio quella citata dagli interroganti, approvata in relazione all'atto del Senato di delega del Governo per la riforma fiscale, che individua nell'ambito della futura attuazione della delega di cui all'articolo 13 un possibile incremento derivante dall'aumento dei canoni di concessione per il gioco *online*. Quanto ai parametri per valutare il giusto livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale, sento comunque di dover precisare che in ogni caso l'incidenza sul PIL è un indicatore ambiguo perché, essendo un rapporto, dipende anche dall'andamento del PIL stesso. Infatti quando si parla della necessità di portare la percentuale del finanziamento corrente sopra il 7 per come è accaduto nel 2020, occorre anche tener conto che in quell'anno il prodotto interno lordo nazionale era crollato di sei punti percentuali, salvo poi risalire negli anni successivi che hanno visto quindi diminuire l'incidenza del finanziamento corrente.

da quello che è un equivoco che viene continuamente raccontato: la percentuale sul PIL, famigerata o fatidica dell'anno del Covid, che evidentemente - essendo la percentuale una frazione di un prodotto interno lordo calato di quasi il 9 per cento in quegli anni anni - dava un risultato più alto. Noi dovremmo semmai parametrare l'attuale percentuale sul PIL alle percentuali degli anni ante Covid che si attestavano intorno al 6

a sistemare nei prossimi cinque-dieci anni il livello di finanziamento del nostro fondo sanitario nazionale che reputo essere indispensabile per mantenere la nostra sanità in linea con le sfide e le richieste di cure che vengono dalla nostra cittadinanza. *(Applausi)*.

dell'egregio signor Ministro una tematica molto sentita, ossia il fatto che ogni anno in Italia i tumori colpiscono circa 2.500 tra bambini e adolescenti;

costituite in molti casi da genitori che hanno perso i propri figli a causa della malattia, e allo stesso tempo le case farmaceutiche non investono in questo tipo di ricerca perché sui tumori pediatrici non ci sono degli incentivanti profitti. È brutto da dire, ma è così e bisogna anche far conoscere qual è

Ci sono dei benefici che indubbiamente questa legge apporterebbe, tra cui sicuramente l'accelerazione nel campo della ricerca e il fatto che venga costituito un comitato di bioetica nazionale dedicato alle malattie nell'età pediatrica: questo faciliterebbe l'immissione di nuovi farmaci

di tumore, l'osteosarcoma, che aggredisce molto bambini e ragazzi. Se si riuscisse a mobilitare questa legge e ad accelerare i decreti attuativi, magari riusciremmo a fare un passo in avanti

sulle sperimentazioni cliniche, desidero segnalare quanto segue: le disposizioni introdotte con la legge n. 3 del 2018 adeguano alla disciplina italiana la nuova normativa europea prevedono il riordino e la riduzione dei comitati etici. Nello specifico, queste norme prevedono l'istituzione di un centro di coordinamento nazionale di comitati etici territoriali per le sperimentazioni cliniche sui medicinali per uso umano e sui dispositivi medici con funzioni di coordinamento, indirizzo e monitoraggio delle attività di valutazione degli aspetti etici relativi alle sperimentazioni. Prevedono, inoltre, l'individuazione di un numero massimo di quaranta comitati etici territoriali rispetto agli oltre cento esistenti prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina, di cui almeno uno per ogni Regione, e il riconoscimento di tre comitati etici a valenza nazionale, di cui uno riservato alla sperimentazione in ambito pediatrico. I decreti attuativi finalizzati a rendere operativa la nuova disciplina dei comitati etici territoriali sono stati adottati. Infatti, con decreto del Ministro della salute del 27 maggio 2021, è stato ricostituito il centro di coordinamento nazionale dei comitati etici territoriali per le sperimentazioni cliniche sui medicinali per uso umano e sui dispositivi medici, già istituito per un triennio

il terzo istituito presso l'Istituto superiore di sanità e rivolto alle sperimentazioni cliniche degli enti pubblici di ricerca e agli altri enti a carattere nazionale. Con il decreto dello scorso 26 gennaio ho individuato i 40 comitati etici territoriali, come indicato dalla medesima legge delega. Con il decreto del 27 gennaio 2023 ho provveduto a regolamentare la fase transitoria, fino alla completa attuazione del regolamento europeo sulla sperimentazione clinica dei medicinali. Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il decreto del 30 gennaio 2023, abbiamo determinato la tariffa unica a carico del promotore della sperimentazione, da applicare in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, stabilito le modalità di versamento della stessa e definito l'importo del gettone di presenza e l'eventuale rimborso delle spese di viaggio per i partecipanti alle riunioni dei comitati etici. Con il decreto del 30 gennaio 2023 ho provveduto poi ad armonizzare la disciplina già in vigore in materia di sperimentazioni cliniche con quanto disposto dal medesimo articolo 2. In particolare sono state definite le funzioni dei comitati etici, i criteri per il riparto delle competenze tra i comitati etici territoriali e quelli a valenza nazionale, nonché i criteri per la loro composizione. Alla luce di quanto rappresentato, posso confermare che, entro gli ambiti della cornice normativa costituita dai decreti ora ricordati, l'Aifa, le Regioni e il centro di coordinamento nazionale dei comitati etici procedono ad espletare le attività necessarie per garantire la piena operatività sia dei comitati etici territoriali di nuova istituzione, sia del sistema nel suo complesso. Per il profilo specifico degli interroganti, faccio presente che il comitato etico nazionale per la sperimentazione clinica pediatrica è già pienamente operativo, a seguito della nomina dei suoi componenti, avvenuta con decreto del 22 marzo 2022 e attivo sia sul portale dell'Osservatorio nazionale sperimentazione clinica, sia sul portale europeo Clinical trials information system. intervenire in replica il senatore Romeo, l'allora Ministro della salute, proprio per sapere a che punto erano i decreti attuativi. Si diceva che c'erano ancora alcuni elementi in fase di istruttoria, che dovevano poi essere resi operativi. Ci fa piacere sapere che il comitato di bioetica nazionale, che si occupa

Signora Presidente, signor Ministro, colleghi, nonostante le gravi carenze di personale, soprattutto per alcune professioni, come quella infermieristica, e nonostante il numero di posti letto sia ben al di sotto della media europea, secondo i dati più recenti dell'OCSE, l'Italia si colloca ben al di sopra della media europea della media europea in termini di esiti clinici, segno di un sistema sanitario nazionale resiliente, che rappresenta ancora oggi, nonostante tutto, un modello di tutela della salute nel mondo. Signor Ministro, di questo dobbiamo tutti andar fieri. Tuttavia, in questo contesto, desta particolare preoccupazione che nel Documento di economia e finanza si preveda una graduale riduzione del Fondo sanitario nazionale, che arriverà a toccare quota 6,2 per cento rispetto al PIL, nel 2025. Ciò rappresenta un ritorno indietro rispetto alle percentuali raggiunte nel 2020, nel 2021 e nel 2022,

Oltretutto, ci tengo a ricordare che i tetti di spesa per il personale sanitario sono stati messi dal Governo Berlusconi, di cui l'attuale *premier* Meloni era Ministro nel 2011, e da allora non sono mai stati tolti, se non alleggeriti, prima dal ministro Madia e successivamente dal ministro Speranza. Voglio ricordare anche che, durante la pandemia, tutti, ma proprio tutti, anche coloro che allora stavano all'opposizione, dicevano di aver imparato la lezione.

oggi lo ha ripetuto - nei giorni scorsi ha dichiarato che sarebbero necessari 3-4 miliardi in più e, siccome il 25 luglio scorso anche il Senato ha approvato una mozione che lo impegnava in tal senso, ci stiamo chiedendo, se davvero lei riuscirà a trovare queste risorse. Siamo contenti, Ministro, che, anziché ripetere, come avete fatto per tutto questo anno - e come ha fatto lo stesso senatore Zaffini poco fa - che non avete definanziato il Sistema sanitario nazionale, ora stiate dicendo che servono altre risorse: siamo felici che ve ne siate accorti, ma siamo preoccupati

Nel corso di oltre un decennio il livello del fabbisogno sanitario nazionale *standard* ha registrato periodi di effettivi tagli, soprattutto in conseguenza delle manovre di *spending review* che sono state adottate anche nel settore sanitario e delle complessive manovre di finanza pubblica, salvo il picco registratosi nell'anno 2020, in corrispondenza degli effetti della pandemia Covid-19. Riguardo ai parametri per valutare il giusto livello di finanziamento del sistema sanitario nazionale ho anche già osservato che in ogni caso l'incidenza sul PIL è un indicatore ambiguo: essendo un rapporto, dipende anche dall'andamento del PIL stesso. Quando si parla della necessità di portare la percentuale del finanziamento corrente sopra il 7 per cento del PIL, occorre anche tener conto che in quell'anno il prodotto interno lordo nazionale era crollato di tanti punti percentuali, salvo poi risalire con vigore successivamente. Altrettanto mi suggeriscono gli economisti riguardo ai dati OCSE: è infatti vero che l'Italia spende meno di Francia e Germania per la sanità, ma il paragone non è sempre corretto. Se Germania e Francia spendono rispettivamente 3.450 e 3.071 euro *pro capite* rispetto ai 2.178 euro dell'Italia per la sanità pubblica nel 2019 è perché la loro economia è più sviluppata e il loro PIL supera quello italiano del 39 e del 20 per cento (la fonte è Eurostat). Ciò vale anche per i redditi dei medici, degli insegnanti e del personale sanitario. L'Italia raggiungerà queste cifre, se e quando il suo PIL toccherà i 35.000-40.000 euro *pro capite*. Inoltre, occorre considerare che l'Italia spende 3,9 punti di PIL più della Germania e 0,4 più della Francia per le pensioni. Abbiamo poi un vincolo pesante, vale a dire gli interessi sul nostro enorme debito pubblico (80 miliardi all'anno) che assorbono l'8,5 per cento della spesa pubblica o il 4,1 del PIL. Mentre la Germania spende solo lo 0,9, la Francia l'1,6 del PIL. In totale sono 6,6 punti di PIL più della Germania e 2,4 più della Francia. Se non ci fossero queste distorsioni, la sanità italiana potrebbe beneficiare di almeno 45 miliardi di euro in più. Da ultimo, per quanto concerne la necessità di incrementare l'organico medico e infermieristico, devo evidenziare che purtroppo il reiterarsi nel tempo delle misure di contenimento della spesa per il personale ha determinato negli ultimi anni una significativa riduzione del personale del sistema sanitario nazionale. Questa situazione, però, soprattutto per la prevalenza del Covid-19, ha ulteriormente acuito le difficoltà del sistema, anche se i dati più recenti, fortunatamente, mostrano una ripresa della numerosità del personale con rapporto di lavoro subordinato. Al riguardo dell'analisi dei dati disponibili è emerso tuttavia che le difficoltà di reclutamento dei professionisti, in particolare di medici ed infermieri, sono determinate non soltanto dai vincoli di spesa ma anche dalla scarsa attrattività del nostro sistema per i professionisti, con la conseguenza che spesso i concorsi non consentono la copertura dei posti per carenza di aspiranti. È pertanto chiara la consapevolezza della necessità di agire in maniera strutturale, sia assicurando le necessarie risorse al sistema, sia migliorando l'organizzazione dei servizi. Nell'ambito della manovra finanziaria che sarà operata con la legge di bilancio 2024 si renderà necessario, pertanto, cercare di reperire apposite risorse per finanziare strumenti incentivanti da destinare al personale del sistema sanitario nazionale e soprattutto al miglioramento del servizio reso ai cittadini. Penso in particolare all'abbattimento dei tempi delle liste d'attesa. Confermo quanto dichiarato nell'intervista richiamata dagli interroganti circa la necessità di destinare maggiori risorse alla sanità e a tal fine rappresento che sono stati avviati tutti gli approfondimenti tecnici per individuare le misure più opportune nell'ambito degli istituti normativi e contrattuali vigenti, fermo restando che le stesse dovranno essere necessariamente concertate con il Ministero dell'economia e delle

dicendo che il problema sta nel passato, mentre il problema, signor Ministro, sta in questo presente che voi non siete in grado in alcun modo di affrontare. È ormai trascorso un anno da quando questa maggioranza è al Governo e noi continuiamo a sentire che è colpa di chi c'era prima. Bisogna evitare che il Servizio sanitario nazionale entri in una crisi che non ha più possibilità di ritorno e noi stiamo arrivando a questo punto. Voi siete al Governo per trovare soluzioni e per cercare davvero una risposta ai bisogni dei cittadini. Le risorse indubbiamente sono in testa a tutto questo, ma occorre anche molto altro, a cominciare dal recupero di un rapporto di fiducia con tutto il personale sanitario, che non ne può più e che è sotto una pressione indicibile. Il Servizio sanitario nazionale, che quest'anno celebra i suoi si basa su tre principi: uguaglianza, equità e universalità. Ebbene, questi tre principi sono tutti messi in discussione dall'avanzare di una crisi che questo Governo non sembra neppure più intenzionato ad affrontare. Noi ci domandiamo che fine abbiano fatto, per esempio, i finanziamenti del PNRR, ma ci domandiamo anche come pensate di affrontare con l'autonomia differenziata il venir meno di questi tre principi che, come dicevo e come ormai ogni dato conferma, vedono l'Italia in una condizione di disparità assolutamente inaccettabile. L'autonomia differenziata e il taglio delle case di comunità produrranno ulteriori danni. Questo ci preoccupa molto. Ci vuole una visione d'insieme che noi non sentiamo in alcun modo avanzare e ci vuole una riforma strutturale, un'azione strutturale, non una ricerca disperata eventualmente di qualche euro in più che comunque sarebbe il benvenuto.

con altri fondi per circa 20,23 miliardi nel periodo 2021-2026; che la componente 1, reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale, ha previsto la realizzazione di 600 centrali operative, 1350 case di comunità per 2 miliardi di euro e 400 ospedali di comunità; che la Corte dei conti, al 31 marzo 2023, ha rilevato che ci sono realistiche difficoltà di pervenire nei tempi ormai ravvicinati al *target* del 31 marzo 2023

previste case di comunità e delle centrali operative; che, a fine 2022, di queste erano complessivamente attive, tra case di comunità, ospedali di comunità e centrali operative, una percentuale minima tra l'8,5 e il 27,8 Inoltre, la relazione sul PNRR, aggiornata al 31 luglio 2023, presenta criticità per eventi e circostanze oggettive che riguardano le case di comunità e gli ospedali di comunità. Citiamo l'aumento dei prezzi delle materie prime ed energetiche, che ha comportato un aumento del costo degli investimenti programmati, soprattutto per le opere di edilizia sanitaria. Tra l'altro, tale evoluzione del contesto delle case di comunità ha portato ad una stima di incremento 24 fino al 66 per cento circa in base alle Regioni considerate, comportando poi la richiesta di questo Governo di una rimodulazione del numero delle strutture realizzabili: per le case di comunità, fino a scendere da 1.350 a 936; per gli ospedali di comunità, da 400 a 304; per le centrali operative, da 600 a 524. Alla luce dei dati appena citati e visti

per reperire le ulteriori risorse necessarie per la realizzazione di tutte le strutture originariamente previste e nei tempi previsti.

Come noto, il Governo in adempimento della risoluzione approvata dal Parlamento il 1° agosto scorso ha provveduto ad inviare la proposta di revisione del PNRR, comprensiva del capitolo REPowerEU, alla Commissione europea e ad avviare le prime interlocuzioni in ordine alle modalità e ai termini per l'attuazione dei successivi adempimenti. La proposta di revisione del PNRR riguarda 144 misure di investimento e di riforma; si compone sia di modifiche formali, mirate ad agevolare la rendicontazione di obiettivi e traguardi, che di modifiche sostanziali, dovute al mutato contesto internazionale, che ha determinato ostacoli oggettivi al raggiungimento di obiettivi e traguardi. Inoltre, si prevede la riallocazione delle risorse verso impieghi più efficienti, che conducano lo spostamento di alcune misure del PNRR ad altre forme di finanziamento. Faccio presente, comunque, che la proposta di revisione e aggiornamento per la missione 6 salute non modifica la dotazione finanziaria complessiva. In realtà la revisione mira a rafforzare l'ambizione della missione, attraverso un uso più efficace ed efficiente delle risorse destinate all'edilizia sanitaria dall'articolo 20 della legge n. 67 del 1988, anche al fine di coprire l'incremento dei costi registrato, stimato in circa il 30 Considerato, infatti, che, a fronte di uno stanziamento pari a 24 miliardi di euro per gli adempimenti correlati all'edilizia sanitaria, risultano programmati solo 14 miliardi circa, la proposta mira ad accelerare l'impiego delle risorse per garantire tutti gli impegni assunti dal nostro Paese con il PNRR. L'impiego di queste risorse nell'ambito del PNRR assicura, inoltre, la realizzazione di tutti i progetti previsti, che, senza questo intervento, rischiavano di non essere realizzati per l'incremento dei costi. La proposta di revisione prevede l'utilizzo delle economie registrate nell'ambito della componente 2 innovazione, ricerca, digitalizzazione del Servizio sanitario nazionale per nuovi interventi che mirano a rafforzare la dotazione tecnologica delle strutture sanitarie. Preciso al riguardo che, per garantire la copertura dei quadri economici dei progetti candidati a valere sul PNRR e di competenza del Ministero della salute, la proposta prevede una rimodulazione dei *target* realizzativi sulle linee di intervento PNRR per controbilanciare l'effetto derivato dall'aumento dei costi dovuti all'innalzamento dei prezzi regionali, all'inflazione, impiegando fondi alternativi alternativi quali quelli correlati agli accordi di programma stipulati con le Regioni dagli interventi previsti dall'articolo 20 ed eventuali risorse derivate da fondi per le politiche di coesione. Comunque, nelle more della finalizzazione delle proposte di rinegoziazione del PNRR, gli uffici preposti garantiscono le attività relative alle istanze per l'ottenimento delle risorse addizionali dal cosiddetto fondo opere indifferibili per gli anni 2022-2023, istituito per fronteggiare l'eccezionale aumento dei materiali da costruzione negli appalti pubblici, nonché le attività di presidio e vigilanza delle realizzazioni, istruendo le richieste di modifica e integrazione del finanziamento PNRR dei progetti con risorse derivanti dal bilancio dei soggetti attuatori. Concludo segnalando che dal puntuale monitoraggio semestrale condotto da Agenas, allo stato non rileva alcuna ragionevole preoccupazione riguardo al rischio che la costruzione ed attivazione delle case ed ospedali di comunità previsti dal PNRR possano non essere completate entro la data stabilita del 30 giugno 2026, come da *target* sulla missione 6. *(M5S)*. Signora Ministro, purtroppo non posso dirmi soddisfatta della sua risposta, anche se avrei voluto sentire parole di novità da lei. Attingere ai fondi dell'articolo 20 per sopperire a quello che non si riesce a fare con i fondi del PNRR è un grave problema, perché quei fondi erano previsti per farci altro. Quindi, se li mettiamo sul PNRR, non ci facciamo le altre cose che avremmo dovuto fare. *(Applausi)*. E non stiamo parlando di campi da bocce; stiamo parlando di ospedali necessari al territorio, perché - come diceva prima la collega Zambito - siamo anche in carenza di posti letto ospedalieri rispetto alla media europea. Abbiamo visto, durante il Covid, quanto riduzione del numero dei posti letto nei nostri ospedali abbia fatto male al nostro Paese. Andavano potenziate la medicina territoriale, con gli interventi del PNRR, e le strutture ospedaliere, con i fondi dell'articolo 20. Invece qui facciamo il gioco delle tre carte, senza arrivare a niente. Oltretutto, non vorrei che poi ci diceste, in separata sede, che gli ospedali invece li realizziamo con i partenariati pubblico-privato, che hanno già manifestato grandissime criticità. Arrivo dal Piemonte, dove stiamo ancora aspettando la realizzazione della città della salute di Torino con il partenariato pubblico-privato, perché i costi sono saliti alle stelle; idem dicasi per quella di Novara. Adesso c'è sul piatto il nuovo ospedale di Cuneo, che presenta le stesse criticità, perché, invece di usare le risorse che ci sono nell'articolo 20, si vuole ricorrere ai finanziamenti dei privati, così alla fine gli ospedali li pagheremo due volte. Mi spiace, ma non ci siamo proprio.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

Non ho chiesto di intervenire prima per rispetto dei colleghi e per la presenza della diretta televisiva, ma ritengo inaccettabile che il Ministro degli affari esteri, nel fornire peraltro una risposta ad un altro interrogante, decida di fare dell'ironia circa la presenza o meno di un senatore all'interno di quest'Aula, considerando il fatto che comunque il Gruppo del senatore cui lui stava facendo riferimento è stato regolarmente presente per tutta la durata Il Gruppo di Azione-ItaliaViva-RenewEuropeinfatti è stato fedelmente presente all'interno dell'Aula del Senato. Se volessimo scendere sul piano del bieco qualunquismo, così come ha fatto il Ministro, potremmo dire che lui stesso

altri colleghi. Credo che questo debba essere stigmatizzato, perché qualunque Ministro che interviene in quest'Aula ha il dovere di portare rispetto a qualsiasi componente del Parlamento, in quanto espressione della sovranità popolare.